Comunico che in data 8 aprile 2021 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»

nazionale. Avverto che è stato altresì presentato l'ordine del giorno G1, dei senatori Binetti, Boldrini, Castellone, Giuseppe, Pirro, Fregolent, Cantù, Zaffini, Parente, Siclari, Iori, Richetti e altri, il cui testo è in distribuzione.

Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, questo periodo, dal punto di vista della storia della medicina, passerà alle cronache come il momento in cui siamo stati capaci di introdurre una nuova classificazione: tra pazienti Covid e gli altri. Devo dire che proprio questo riduzionismo semantico ha comportato, però, conseguenze molto gravi in quella che è la vita di moltissimi pazienti

A mio avviso sono errori strutturali il cui prezzo più alto lo pagheranno i pazienti. La nostra mozione in qualche modo ripercorrere queste tappe, che sono quelle tipiche per cui è stato possibile negli anni permettere che tutta l'oncologia facesse passi avanti da gigante. Concretamente, anche in Italia sono molti i centri di oncologia di assoluta eccellenza. L'oncologia ha potuto fare passi avanti per ragioni molto chiare: la prima è che siamo stati capaci di concentrarci su *screening* precoci che hanno permesso diagnosi quando il tumore era ancora alle sue prime battute. Ebbene, quello che è accaduto in questo periodo è che c'è stato uno *stop* agli *screening* che ha rallentato se non proprio la diagnosi, perlomeno il sospetto della diagnosi. Certamente, infatti, dopo una prima diagnosi emersa dallo *screening*, si passa a un approfondimento diagnostico che richiede strumenti più sofisticati, metodiche di *imaging*, strumenti di laboratorio, indagini molto più complesse che permettono di arrivare a

Di tutto questo, in questo lungo anno di *lockdown*, possiamo dire che c'è stato davvero molto poco e le conseguenze di tutto ciò le pagheremo nel tempo, perché i casi che non abbiamo diagnosticato oggi esploderanno tra qualche giorno. Avremo forse vinto la battaglia dei vaccini, cosa che ci auguriamo, ma avremo perso la battaglia su questi altri fronti. Richiedere con insistenza e con energia un nuovo Piano oncologico

della medicina italiana. Pertanto, il paziente con una maggiore disponibilità economica ha potuto fare riferimento a strutture private, in cui fare gli approfondimenti necessari, ma questo si è convertito in un ulteriore fattore di discriminazione tra chi può e chi non può, mentre noi riteniamo la salute un bene uguale per tutti, che va difeso nello stesso modo per tutti.

*ad integrum*, ovvero alla loro vita normale. Tutto questo è venuto meno e di tutto questo siamo responsabili anche noi. A tutto questo dobbiamo mettere un freno e dobbiamo ripartire nel miglior modo possibile. *(Applausi)*.

Binetti - è importante perché rafforza gli intenti del Parlamento nei confronti del Governo. Ci siamo resi conto in effetti anche in questa emergenza che soprattutto per i malati oncologici persiste una grave e inaccettabile diseguaglianza territoriale e quindi la presa in carico dei pazienti, anche in questo caso, purtroppo non è omogenea. Questo è il motivo per cui anche oggi noi tratteremo un tema così importante: la mancata integrazione, di cui purtroppo ci rendiamo conto, tra ospedale e territorio rappresenta ancora oggi uno dei più grandi *deficit* organizzativi del Servizio sanitario nazionale.

Sappiamo che gli strumenti per poter attuare le linee guida sono essenziali e fondamentali. Il fatto di avere a disposizione

dobbiamo attuare altri protocolli che possano dare un aiuto importante anche ai nostri professionisti. Ritengo non meno importante, come sottolineo sempre, l'adozione di iniziative volte a garantire

rafforziamo ancor di più il sistema per i professionisti che ne hanno necessità, ma soprattutto per i nostri malati che stanno attendendo che ci siano delle indicazioni particolari omogenee per tutto il territorio nazionale. Dichiaro quindi sin da ora che ritirerò la mia mozione per farla confluire in un ordine del giorno unitario. Ringrazio

abbiamo voluto che gli impegni contenuti nelle nostre mozioni convergessero in un unico strumento affinché esso potesse avere la forza di incidere proprio a livello governativo. Ci auguriamo che questo lungo lavoro fatto tra di noi per cercare il punto di vista unitario, attraverso il confronto che c'è stato, pesando la responsabilità che ad ognuno degli impegni viene legata affinché si garantisca un diritto reale da parte dei pazienti...

voglio ripartire da questo punto. Noi sappiamo bene che un ordine del giorno è uno strumento debole sotto il profilo normativo,

La forza del documento risiede nel fatto che tutto il Senato si schiera dalla parte dei malati oncologici, ne riprende e ne pone in *pole position* il diritto alla cura, prima il diritto alla diagnosi, poi il diritto ad essere integrato in un progetto fortemente personalizzato, che risponda anche all'evoluzione della scienza e della tecnica. Ma la forza dell'intero Senato non potrà giustificare nessuna elusione di responsabilità. Per fare un esempio, signora Presidente e dirlo ai colleghi, uno dei passaggi è quello per cui noi chiediamo la piena attuazione di una legge che abbiamo approvato due anni fa.

inattuata e oggi potrebbe risultare invece preziosissima per riorientare il lavoro, anche nella direzione suggerita dalla collega Boldrini, cioè quella di ridurre le discriminazioni sul piano nazionale: offrire a tutti i malati gli stessi diritti, lo stesso accesso alla diagnosi, lo stesso accesso alla terapia stesso accesso a una riabilitazione sociale. Un piano nazionale è fondamentale: due anni fa il Parlamento ha approvato una legge che però non è operativa. L'ordine del giorno presentato oggi intende "graffiare" questo anonimato delle richieste che, anche se approvate, cadono in sacco vuoto. noi siamo tutti impegnati e l'intera Commissione, nell'arco di quel che resta di questa legislatura, si batterà perché ognuno di questi impegni che abbiamo sottoposto al Governo

Noi abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo superato le nostre diversità di opinioni, i nostri gusti personali, le priorità con cui si potevano segnare una cosa e l'altra; abbiamo deciso che veramente uniti si poteva vincere questa battaglia. È una sfida che assumiamo come un valore straordinario, a garanzia dei diritti dei malati, in particolare oggi dei malati oncologici. Signor Presidente, rappresentanti che tutti noi portiamo sulla nostra pelle lo stigma della malattia oncologica, o perché in molti casi ha colpito noi stessi o una persona cara, o perché ha colpito o potrebbe colpire qualcuno che ci è molto vicino. Questi malati ci guardano negli occhi e ci chiedono con quale coraggio possiamo dimenticarci di loro, di quella che molte volte è stata soprannominata la malattia del secolo. secolo. Oggi l'oncologia rappresenta una miniera d'informazioni scientifiche, di possibilità di sperimentazione. Vorrei dire una cosa che ritengo sarà abbastanza interessante anche dopo, quando si discuterà la mozione sui vaccini. Il miracolo - perché tale è stato definito - del vaccino, concretamente di quelli di Pfizer e Moderna, è stato possibile perché quel gruppo di studiosi stava studiando meccanismi di azione e terapeutici che riguardavano i tumori; stavano studiando le terapie gli anticorpi monoclonali e hanno avuto l'intuizione di applicare al *virus* un meccanismo di studio che fino a quel momento era stato dedicato al tumore. La scienza ha questa potenza traslazionale che garantisce a tutti che il diritto alla salute non sia solo una semplice parola, ma sia un fatto concreto che impegna tutti noi davvero a garanzia di un bene straordinario, di un diritto straordinario. *(Applausi)*.

supera qualunque plausibilità delle singole mozioni.

Signor Presidente, cari colleghi, care colleghe, in questo anno e mezzo molte persone hanno dovuto fare i conti con le ripercussioni della pandemia sul Sistema sanitario, con interventi chirurgici rinviati, esami e visite specialistiche cancellati, reparti ospedalieri che non hanno potuto far fronte alla normale attività quotidiana. Si tratta di una sorta di epidemia nell'epidemia, che ha coinvolto migliaia di pazienti che hanno contratto neoplasie, malattie oncologiche proprio nell'anno più drammatico che la sanità abbia dovuto affrontare. I recenti dati diffusi da Agenas indicano la dimensione di questo dramma. Nel corso della pandemia, sono andati perduti 52 milioni di visite specialistiche e prestazioni diagnostiche,

di interventi per il cancro al seno, il 24 per cento in meno di interventi per il cancro alla prostata e il 32 per cento in meno per il cancro al colon. In Lombardia, una delle Regioni più colpite, ma anche una delle Regioni che ha i centri migliori per i tumori, i numeri sono ancora più gravi e questo fa riflettere. L'epidemia di Covid ha messo a dura prova la capacità di risposta e di resilienza dei sistemi sanitari a livello regionale, mettendo a rischio il lavoro di prevenzione e controllo dei tumori, che è lo strumento primo che abbiamo a disposizione per combatterli. In questo quadro, le disuguaglianze si sono allargate, creando un solco sempre più profondo tra le persone abbienti o con un più alto livello di istruzione, che hanno potuto ricorrere alla sanità privata, e i più fragili, che non hanno potuto accedere ai percorsi di *screening* pubblici. Si tratta di un fatto grave, con cui dovremo fare i conti, perché si tratta di un *vulnus* che mi auguro sarà sanato con la nuova ripresa impressa al piano vaccinale. Il primo obiettivo, dunque, è mettere in campo una strategia per ripristinare in tempi rapidi quantomeno il livello di assistenza per i malati oncologici garantito prima della pandemia, perché il Covid è arrivato come uno *tsunami* su un sistema che mostrava già delle carenze strutturali e dei ritardi nell'adeguamento tecnologico del Servizio sanitario nazionale in ambito oncologico. Un sistema in cui vi sono enormi differenze territoriali, differenze che l'epidemia non ha fatto che ampliare. Pensiamo, ad esempio, alla telemedicina, che sarà una delle chiavi della sanità del futuro, il cui sviluppo è legato alla digitalizzazione dei servizi e alla diffusione dell'innovazione. Proprio la telemedicina offre infatti la cifra della grande variabilità territoriale anche nell'ambito del servizio sanitario regionale. Nei prossimi mesi, dunque, dovremo compiere il massimo sforzo per ridare speranza ai vulnerabili e in particolare per quanto riguarda i pazienti oncologici bisognerà agire in fretta, intervenire subito. Dobbiamo quindi perseguire questo impegno comune, ovvero migliorare l'assistenza dei malati oncologici attraverso un nuovo Piano nazionale il potenziamento delle reti territoriali, la promozione degli *screening*, il rafforzamento dell'assistenza domiciliare, la modernizzazione della dotazione strumentale e tecnologica per gli *screening* diagnostici, per le attività chirurgiche, per la radioterapia; potenziamento della sanità digitale, gli investimenti nella ricerca per il sostegno psicologico ai malati oncologici, come previsto dai LEA. questi pazienti e le loro famiglie, oltre che delle cure sanitarie, hanno bisogno di un supporto emotivo costante, che contenga anche il dolore dell'anima e la fragilità di dover affrontare una malattia che mette a rischio la vita e prevede terapie dolorose da tutti i punti di vista. Occorre quindi investire sull'assistenza territoriale, perché solo un'idea comunitaria di sanità riuscirà a garantire a tutte le persone di affrontare la malattia oncologica con percorsi che tengano conto dei loro bisogni di salute.

Signor Presidente, non si capisce come mai le preoccupazioni e le virtù siano esplose solamente dopo una pandemia che non perdona. Oggi siamo qui a discutere la mozione sull'adozione di un nuovo piano oncologico, scaduto già nel 2016, pubblicato nel 2013 ed elaborato almeno cinque anni prima: è paradossale. Lo stesso è accaduto per il piano pandemico e chissà per quante altre gravi patologie. Eppure, i pazienti oncologici devono poter beneficiare di ogni possibile strumento, così come i pazienti affetti da altre patologie. Ora ci si fa paladini di iniziative che avrebbero dovuto essere attuate ed elaborate prima della data di scadenza e non, come in questo caso, cinque anni dopo. Ora si scopre addirittura che i pazienti oncologici e i pazienti con altre gravissime cronicità, oltre al problema per la sopravvivenza, hanno anche altri due gravi problemi: quello economico - e non voglio nemmeno pensare che ci sia qualcuno che abbia dei dubbi al riguardo - e quello psicologico che, intuitivamente, esordisce in concomitanza alla diagnosi. scatta alle giovani madri colpite da questo flagello è il seguente: se non dovessi farcela, chi si prenderà cura del mio bambino? Vi parlo ovviamente per esperienza personale. personale. Esiste anche un terzo problema che sembra sempre sfuggire, quello psichiatrico, quello delle allucinazioni uditive, visive e sensoriali, perché il tumore non è un fattore protettivo per la schizofrenia o per gli altri disturbi mentali. Anche i pazienti psichiatrici si ammalano di cancro. Quindi, cerchiamo di uscire dai muri ideologici e rendiamoci consapevoli di questa realtà, di tutte le conseguenze derivate e dei limiti imposti. È chiaro che sono stati commessi gravissimi errori. Detto ciò, preferisco guardare al futuro. Abbiamo un intero Sistema sanitario da risollevare e da sviluppare in funzione dei progressi tecnologici e scientifici, adottando adottando e promuovendo nuovi modelli, stanziando risorse necessarie per incentivare iniziative strategiche che vadano oltre il modello animale, dove il povero topino e altre creature hanno già dato tutto ciò che potevano dare. Si deve cambiare paradigma; se non si adottano avanzati protocolli di calcolo ad alta prestazione, ponendo le basi per una ricerca innovativa e proficua, si continuerà a inciampare sullo stesso gradino. Nel settore di astrofisica - per esempio - nel cui ambito gli scienziati non hanno nemmeno il materiale da manipolare e possono osservare solo attraverso una lente, a milioni di anni luce, la straordinaria e creativa intelligenza umana era già su Marte prima ancora di partire. In tal senso, vi dirò con grande orgoglio nella mia virtuosa Regione una *startup* creata da tre giovanissime eccellenze ha messo al servizio della diagnosi precoce la propria scienza ingegneristica, dal Polo tecnologico al Centro di riferimento oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone, creando un *software* composto da algoritmi in grado di interpretare in modo oggettivo i tumori ovarici. In questa innovativa e attuale direzione si sta muovendo la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste Magia? No: espandere e scoprire i nuovi mondi, micro e macro, dal pianeta alla proteina, richiede intuizione ed eccellente competenza. che questa mozione sia solo una *ouverture* alla consapevolezza che tutti noi dobbiamo avere per agire tutti insieme, di concerto e in sinfonia, così come è possibile fare oggi. Grazie per l'attenzione colleghi. membri del Governo, onorevoli colleghi e colleghe, la lotta al cancro rappresenta uno degli obiettivi più audaci e stimolanti per il mondo intero, per l'Europa e per il nostro Paese. La ricerca, la diagnosi precoce, i programmi di *screening* diagnostici, il miglioramento dell'approccio multidisciplinare di alta specialità, la disponibilità e la diffusione delle nuove terapie come quelle con l'identificazione di strutture adeguate con la presenza di personale altamente specializzato e gli opportuni percorsi di *follow-up* per i malati di cancro devono rappresentare una necessità e un obbligo delle istituzioni nei confronti dei cittadini. L'obiettivo della missione europea con il nuovo piano oncologico è ben rappresentato dallo *slogan* «*Cancer: mission possible*», il cui obiettivo è salvare, entro il 2030, 3 milioni di vite umane. La grave crisi globale che la pandemia comportato ha avuto importanti e potremmo dire drammatiche ripercussioni su tutta l'assistenza sanitaria, coinvolgendo tutte le patologie che potremmo definire no-Covid, con particolare riguardo alla patologia neoplastica. Risorse economiche importanti non più disponibili, riorganizzazioni strutturali e di personale, la necessità di riconvertire l'utilizzo e la destinazione di intere unità operative ospedaliere dirottate verso la patologia Covid hanno comportato e comportano gravi conseguenze negative sui programmi di prevenzione, assistenza e *follow-up* dei pazienti con altre patologie, in particolare quelli con tumore. Diagnosi, interventi e cure ritardate in molti centri oncologici hanno purtroppo rappresentato quasi la *routine* durante questa terribile pandemia. Si è ridotto il numero di interventi chirurgici, così come - d'altronde - molte sedute di chemio e radioterapia sono state rinviate. Queste affermazioni scaturiscono da dati oggettivi facilmente recuperabili e drammaticamente sono divenute quasi una *routine* nelle nostre strutture sanitarie (anche in quelle di eccellenza). L'incidenza e il peso della grave situazione che stiamo vivendo hanno stravolto l'organizzazione di molti ospedali e dei loro centri oncologici, soprattutto nei Paesi e nelle Regioni economicamente più deboli, in cui la situazione sanitaria sia organizzativa, che strutturale pre-pandemia era già molto carente e nei quali il SARS-CoV-2 ha letteralmente stravolto la loro debole rete oncologica, la cui sopravvivenza, indispensabile anche per il *follow-up* successivo dei pazienti seguiti, si reggeva spesso sui mille sacrifici e sulla lodevole abnegazione dei tanti operatori sanitari. Proprio questi ultimi sono stati spesso trasferiti nelle reparti Covid dedicati, distogliendo una risorsa importante dai difficili equilibri esistenti nei reparti di oncologia. Ad aggravare ulteriormente la situazione si aggiunge che una parte importante delle risorse economiche disponibili è stata dirottata verso l'emergenza sanitaria pandemica, con tagli cospicui ai finanziamenti riduzione dei posti letto e del personale, fino alla chiusura di interi reparti e alla loro riconversione. È stato già detto che - come era logico supporre - i Paesi e le Regioni a basso reddito pagano per tutto ciò il prezzo più alto in termini di qualità di assistenza e di quantità delle prestazioni erogate e, purtroppo, di vite umane. La pandemia ha reso più difficile ottenere cure di qualità e di continuità assistenziale non solo nel campo della patologia oncologica. Da qui la necessità di provvedere con urgenza a un nuovo Piano oncologico nazionale coordinato al piano europeo. Esso deve porre al centro della programmazione le reti oncologiche regionali, collegate alla più vasta rete nazionale, con una vera e propria cabina di regia e di monitoraggio specifica per l'oncologia. Occorre potenziare l'assistenza oncologica domiciliare e territoriale nell'ottica di ridurre il numero degli accessi alle strutture ospedaliere, facilitare un *follow-up* più attento e meno traumatizzante, con un accesso semplificato per i pazienti alle forme di riabilitazione socio-sanitaria che consenta loro un inserimento tempestivo nella vita sociale e professionale; tutto ciò senza dimenticare un nuovo impulso ai programmi di *screening* diagnostici. Signor Presidente, sarà importante dare un nuovo *input* e una corretta attenzione alle misure che l'istituzione del registro nazionale dei tumori, approvato da questo Parlamento, ha reso non più differibili e procrastinabili. La pandemia ha reso tutto oggettivamente più difficile, ma non per questo impossibile. È indispensabile, pertanto, fare un'attenta riflessione sui dati e programmare il nuovo Piano oncologico nazionale.

a dispetto del numero di pagine che mi sono state fornite dal Ministero. Devo ringraziare tutti voi per le mozioni, *in primis*, e per l'ordine del giorno che avete presentato. Purtroppo mi trovo a rivivere qualcosa che non è lontano dal piano pandemico. Così come avevamo un piano pandemico molto vecchio, aggiornato, riaggiornato, pubblicato - è un qualcosa che era previsto per l'influenza - per quanto riguarda l'oncologia - e ringrazio la senatrice Binetti - siamo fermi a 2011, con una proroga fino al 2016; e dal 2016 ad oggi, per quanto io possa aver studiato e cercato, non ho trovato nulla fino al 2019. O meglio, vi è una bozza

e chiedo scusa a nome del Ministero. Anche se sia io che il ministro Roberto Speranza siamo lì da poco tempo, sono doverose delle scuse per ognuno di voi e per ogni italiano per gli anni di ritardo. Sarà ovviamente mia premura seguire il nuovo documento e far sì che venga approvato senza dover aspettare altri cinque anni. Voglio sperare che tutto ciò accada con un documento che possa essere inviato alla Conferenza Stato-Regioni entro giugno. entro giugno. Se leggo ciò che mi è stato scritto, ossia «tenuto conto del progredire delle conoscenze scientifiche in materia di oncologia e degli strumenti resi disponibili»,

un'indagine compiuta a livello globale su centri oncologici dice che appena il 12 per cento è riuscito a mantenere i livelli di cura pre-pandemia. In Italia, nel 2020, si sono persi migliaia di esami diagnostici e si è registrato un meno 17 per cento di interventi chirurgici e un meno 14 per cento Con i ritardi accumulati dallo *screening* di massa al seno, che è il principale strumento di prevenzione nella relativa patologia, in questi mesi ci siamo purtroppo persi per strada 2.800 tumori. Tutto questo, nella migliore delle ipotesi, si tradurrà in cure più invasive e più costose e dico nella migliore delle ipotesi, perché c'è il rischio che molte malate non scoprano il tumore per via della stretta affinità tra l'identikit del malato medio e i soggetti più esposti all'attuale crisi economica. La pandemia si è portata via un pezzo della nostra sanità e, nel farlo, ha esposto al pericolo soprattutto i pazienti più deboli e, in particolare, gli oncologici. Dati alla mano, un paziente oncologico che si ammala di Covid raddoppia le proprie criticità di salute. Occorre quindi garantire in tutto il territorio nazionale un rapido ritorno alla normalità sul fronte degli *screening*, delle visite, degli interventi e delle terapie. In questi mesi, in particolare in alcune Regioni, l'unica possibilità per visite post-operatorie è stata offerta dagli ambulatori e dalle strutture private e questo anche perché non si è fatto tutto il necessario per sviluppare - per esempio - la telemedicina e le reti territoriali di assistenza. Ancora oggi in Italia abbiamo difficoltà a introdurre le televisite, quando in altri Paesi si è già livello 2 della sanità a distanza, ossia il telemonitoraggio dei valori dei pazienti che presentano malattie croniche. È ovvio che certamente con la telemedicina non si può sostituire il rapporto medico-paziente, ma può essere di grande aiuto. Sulla medicina generale la pandemia ci ha mostrato quanto siano strategici un suo reale potenziamento e miglioramento, nell'idea che la salute non passi solo dai centri specializzati in eccellenza; anzi, la riconsiderazione e il rilancio della medicina generale è di primaria importanza per garantire l'assistenza alle fasce più deboli, agli anziani e a coloro che vedono nel medico di famiglia un punto di riferimento. Da questo punto di vista bisogna però riflettere, una volta per tutte, su quale è oggi nel 2021 la missione principale dei medici di assistenza primaria. Si tratta di una professione che negli anni è stata sovraccaricata di compiti che si sono stratificati (la diagnosi, la cura, la prevenzione, le vaccinazioni, una montagna di burocrazia), che rischiano di rendere meno efficace o addirittura di paralizzare un servizio che dovrebbe essere invece il perno della sanità territoriale. modo, è arrivata l'ora di integrare realmente l'attività della medicina generale - quindi i medici di famiglia - con gli specialisti ospedalieri, con le professioni sanitarie - penso, in particolare, agli infermieri - per creare quelle aggregazioni sanitarie territoriali veramente innovative, che sappiano diventare il reale filtro e la prima risposta efficace ai bisogni sanitari della popolazione, soprattutto dei malati oncologici. Tutto questo è ancora più vero e necessario nelle aree interne, soprattutto nelle zone di montagna. Tornando a ciò che viene richiesto con la mozione in esame, adottare un Piano oncologico nazionale significa soprattutto farsi carico, non del paziente, ma della persona. Il percorso per la guarigione richiede tempo e sacrifici. La maggior parte dei malati, infatti, capisce presto che si tratta di una malattia con la quale si convive o, meglio, che la si sconfigge non rinunciando completamente alla propria esistenza. Non a caso, sempre di più i malati oncologici riescono a coniugare lavoro e terapie, se l'ambiente di lavoro e il contesto che li circonda permettono loro di combinare con adeguata flessibilità e ragionevoli aggiustamenti tempi di lavoro e cura. Vorrei spendere ancora una parola su un tema a me molto caro, quello della prevenzione primaria, che anche in campo oncologico assume un'importanza strategica: una corretta alimentazione, stili di vita sani, un'adeguata e costante attività fisica contribuiscono a evitare l'insorgenza di tante patologie oncologiche. Sappiamo poi come azioni di prevenzione secondaria come l'attività fisica e l'allenamento sportivo costante possano addirittura essere efficaci quanto una chemioterapia, ad esempio in certi tumori della mammella. Allora è strategico definire come attuare in modo più efficace possibile un grande piano di prevenzione per tutta la popolazione, che coinvolga tutti gli operatori sanitari del territorio e dell'ospedale. Così come è importante, per via anche dell'abbassamento dell'età media di malati, farsi carico di quei pazienti che sono in condizioni di precarietà lavorativa, perché l'incertezza non aiuta di certo i percorsi di guarigione. È dunque importante implementare modelli di *welfare* capaci di creare sinergie fra sanità, previdenza, terzo settore e mercato del lavoro, affinché si generino contesti adeguati ai malati oncologici. Per concludere, è importante farlo adesso: la pandemia ha mostrato limiti e necessita di un Sistema sanitario da rafforzare attorno ai principi dell'universalità delle cure e della prossimità con tutti i cittadini, a cominciare dai più fragili e dai più bisognosi. Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie sull'ordine del giorno comune che è stato presentato.

con lo spirito di verità che spesso contraddistingue il Sottosegretario. Siamo tutti impegnati, il Governo per primo, per avere un nuovo Piano oncologico nazionale, in sinergia con quello europeo che si sta rinnovando. Forse, se dal 2016 avessimo rinnovato il Piano oncologico nazionale nella direzione assunta da questo ordine del giorno, dalla protezione delle cure domiciliari e territoriali allo sviluppo delle cure domiciliari e alla telemedicina, non avremmo avuto l'unica possibilità di andare in ospedale quando siamo pazienti oncologici e quindi probabilmente non avremmo abbandonato le cure di quei pazienti. Purtroppo la natura fa andare avanti le altre malattie - non solo queste - anche quelle cardiopatiche e altre che sono state trascurate. Naturalmente le scuse più grandi vanno in questa direzione, dal momento che abbiamo trascurato e ancora trascuriamo i malati

della strumentazione, dalla radioterapia ad altri strumenti. Bisogna rinnovarli, perché la tecnologia va avanti e ci sono macchine diverse che curano meglio i pazienti.

se non alla guarigione - naturalmente l'auspichiamo per tanti pazienti - almeno alla cronicizzazione del malato oncologico, e questo si fa attraverso la diagnosi precoce. Quanti *screening* stiamo perdendo in questa fase di epidemia non diagnosticando precocemente un tumore? Occorrono una diagnosi precoce, le cure, le terapie innovative - come ha detto molto bene la senatrice Binetti

un circolo virtuoso tra una legge acquisita e i decreti attuativi, che poi spetta al Governo emanare. Troppe sono le lungaggini in questo Paese, e poi ci troviamo con un'epidemia di certe dimensioni

fondamentale l'intervento del Governo e siamo tutti impegnati per l'attuazione in tempi brevi di tale ordine del giorno, che ci accingiamo a votare unitariamente.

si potrebbe riepilogare in una semplice manifestazione di gioia per il fatto di essere favorevoli tutti, emiciclo del Senato, su un provvedimento così importante e fondamentale. Consentitemi, però, una piccola digressione politica. La settimana scorsa abbiamo condiviso un documento che sostanzialmente chiedeva al Ministro, al Ministero e a tutto il

di aggiornare un protocollo per le terapie domiciliari fermo al novembre dello scorso anno, sulla vicenda Covid-19.

all'attività che avrebbero dovuto esperire il Ministro, come vertice della piramide, e il Ministero nella sua interezza, per per aggiornare i protocolli e aderire a una realtà, che è quella dell'emergenza pandemica, che riempie tutti i giorni la vita quotidiana degli italiani. Oggi sostanzialmente ci troviamo a fare una cosa del tutto analoga: per iniziativa della collega Binetti, ma complessivamente a seguito del dibattito che abbiamo svolto in Commissione, ci troviamo a dover sollecitare l'elaborazione di un Piano nazionale dell'oncologia fermo dal 2016. Verosimilmente - come è stato descritto nelle premesse - questo piano sarà stato elaborato, conoscendo i tempi, almeno nei mesi precedenti, se non negli anni precedenti. Quindi, ci troviamo ad affrontare una realtà sulla materia oncologica, rispetto alla quale - come ha detto perfettamente il rappresentante del Governo - quotidianamente intervengono progressi della comunità scientifica assolutamente fondamentali, e a dover operare e sollecitare un piano che giace da sei-sette anni: davvero del tutto incomprensibile! A tutto questo si aggiungono le gravi circostanze che hanno imposto di accantonare

Ad oggi abbiamo sospeso oltre 2 milioni di prestazioni in *follow-up*; abbiamo sospeso un numero rilevantissimo di interventi chirurgici nel contrasto delle patologie oncologiche e soprattutto gran parte dei modelli di *screening* che erano attivati sul territorio.

all'onestà intellettuale - non vedo altro termine - e alla sincerità del rappresentante del Governo, il collega Sileri, con il quale

ci sono provvedimenti attuativi che ritardano da anni, anche nell'emergenza sismica come nell'emergenza pandemica. Quindi, anche laddove esistano

che attiene alle terapie oncologiche, e mi riferisco in particolare all'intero parco delle attrezzature per la radioterapia oncologica. Su questa materia ci sono stati anche dei provvedimenti legislativi, che peraltro hanno circoscritto, con dubbia

sono addirittura scaduti i contratti di manutenzione. Quindi abbiamo delle apparecchiature che, probabilmente, invece che curare, complicano ulteriormente gli effetti collaterali

Signor Presidente, colleghi senatori, l'emergenza Covid ha messo a dura prova gli ospedali e le strutture sanitarie malati di altre patologie, altrettanto gravi, come i malati oncologici, hanno purtroppo smesso di curarsi. La conferma è arrivata anche durante la presentazione di uno studio recentissimo dal Censis, della settimana scorsa,

visto e considerato che la salute della donna ci sta molto a cuore, le circa 2.000 diagnosi in meno di tumore alla mammella. Sapendo che è altissima la percentuale di sopravvivenza nei casi di tumore alla mammella,

qualcosa con cui dovremo fare i conti appena la tensione del Covid si allenterà, ciò che spero avvenga presto. Dovremo allora fare in modo che in fase più avanzata queste neoplasie vengano individuate in maniera più celere.

AIRO, SICO, SIPO) e della FNOPI, hanno predisposto e promosso un documento programmatico condiviso, delineando una strategia per superare l'emergenza COVID-19 e ripristinare, nel più breve tempo possibile, il livello di assistenza per i malati di cancro garantito fino all'inizio

sono stati tenuti in considerazione a livello internazionale ed europeo. Uno degli ambiziosi programmi dell'Horizon Europe vuole rispondere alle grandi sfide sociali a cui adattarsi e ai cambiamenti climatici

tenendo in considerazione tutti gli aggiornamenti di cui parlava il Sottosegretario prima e sapendo che ci sono sempre delle terapie innovative che possono dare ulteriori possibilità ai malati di cancro per avere una vita più longeva,

per gli *screening* diagnostici. Prima si riesce ad individuare il tumore, prima si riesce a combatterlo e anche a sopravvivere. Questi sono quindi impegni importantissimi che noi vogliamo mettere in evidenza. Un'altra attività importante in questo momento di emergenza Covid è continuare a facilitare anche la consegna dei farmaci a domicilio. Era già stato previsto in tanti provvedimenti sul Covid, continuiamo a farlo affinché i nostri pazienti evitino di girare; a questo punto deve girare chi è in buona salute, non chi invece ha bisogno di essere tutelato. Questi sono tutti impegni che noi chiediamo al Governo, insieme a quello non meno importante, come ho detto anche questa mattina in un'audizione che abbiamo fatto in 12a Commissione, del supporto psicologico.

per il lavoro fatto. Noi condividiamo pienamente l'ordine del giorno G1 che ci apprestiamo a votare; ne approfitto per fare solo due riflessioni. Credo non possa essere una sorpresa per nessuno il fatto che la pandemia abbia avuto conseguenze pesantissime sul Sistema sanitario nazionale, che scontava limiti e problemi strutturali precedenti la pandemia Proprio sulle questioni oncologiche, dove vi sono delle sfide decisive, il nostro Paese deve assumere degli orientamenti politici chiari: non basta dire che occorre la medicina territoriale, non basta dire che occorre l'assistenza domiciliare. Bisogna dire come si vuole l'assistenza domiciliare e la medicina territoriale; vogliamo andare nella direzione di rafforzare una *governance* del sistema integrato, e multiprofessionale attraverso i distretti e la *governance* pubblica

erano sostanzialmente sulle malattie oncologiche e su quelle cardiovascolari, perché qui c'è il mercato. qui c'è il mercato. Non è un caso che non abbiamo ancora un vaccino per l'AIDS e abbiamo solo le terapie. Ce lo vogliamo porre questo problema? problema? Se vogliamo fare un salto di qualità, questo è un tema da cui non si può sfuggire. Una terapia oncologica innovativa costa il 2.000 per cento in più di una vecchia terapia oncologica. Come garantiamo l'universalità?

e le conseguenze di trasformazione dell'assetto produttivo del nostro Paese, pensando prima di tutto all'area della pianura padana, dove le conseguenze sono enormi. Non vorrei che semplificassimo, sono giorni tristi quelli nei quali si cerca di trovare un capro espiatorio, capro espiatorio, in cui ciascuno pratica lo sport più diffuso in Italia, che non è il calcio, ma è dare la colpa a qualcun altro. non va bene e non ci convince. Si può fare propaganda, ma non si risolvono i problemi. Per risolvere i problemi ci vuole coesione, ci vuole una visione

prima di tutto il Governo che deve dare esempio di coesione e deve darci una traccia strategica, perché così possiamo affrontare una discussione seria e non scaricare il barile, ma fare un salto di qualità. Penso che abbiamo tanti problemi difficili la risposta più sbagliata è e sarebbe semplificare senza risolvere i nodi fondamentali.

il Governo ci dica quali sono le scelte che propone e ci consenta di fare una discussione seria, alla ricerca di quel salto di qualità che, lo ripeto, si fa solo con la coesione

Signor Presidente, anche per le malattie oncologiche, come è stato ricordato un po' da tutti, durante la pandemia Covid è stato ricordato un po' da tutti, durante la pandemia Covid il nostro Servizio sanitario nazionale ha evidenziato alcune sue criticità e fragilità già presenti, che si sono ovviamente pesantemente aggravate a causa dell'epidemia. Sono stati citati i dati relativi agli *screening* oncologici, quindi alla possibilità di diagnosi precoce in persone sane in quel momento o perlomeno senza sintomi: il ritardo o la carenza di *screening*, evidentemente, ci ha fatto individuare meno tumori. Gli altri li individueremo in futuro, nei prossimi mesi e nei prossimi anni e saranno quasi certamente in uno stadio più avanzato. Quindi, anche se il virus magicamente scomparisse domani, ci porteremmo avanti queste conseguenze della pandemia ancora per diversi anni. Oltre allo *screening*, anche la diagnosi di un tumore deve essere tempestiva. La pandemia ha fatto sì che si allungassero le liste di attesa per vari esami diagnostici necessari per diagnosticare il tumore, oppure per una valutazione preoperatoria, nel caso in cui l'esito fosse la chirurgia. Le liste d'attesa chirurgiche

perché molto facilmente queste persone dovranno subire interventi chirurgici più invasivi, più demolitivi e alla fine più invalidanti. Questo nei casi forse meno sfortunati, perché in molti altri si rischia addirittura di non riuscire ad arrivare in tempo. Poi, c'è tutto quello che viene dopo l'intervento chirurgico, quando necessario, come la riabilitazione. In epoca Covid, i reparti di riabilitazione sono stati convertiti in reparti Covid per accogliere tali

E pensare che la scienza fa continuamente progressi enormi nella terapia dei tumori, che cambia ed evolve costantemente costantemente e la medicina di precisione è sempre più personalizzata. L'importante però è che le persone riescano ad avere accesso a queste cure. L'attuale

croniche, con cui una persona può convivere abbastanza bene, spesso con una qualità di vita buona anche per numerosi anni. Quindi, un sistema sanitario che dedica sempre più attenzione alla cronicità, vista anche la situazione demografica del nostro Paese, deve deve rivolgersi in modo importante alla cura e al trattamento di queste patologie.

la necessità di controllo, di monitoraggio e di coordinamento di tutto questo. Un altro versante dell'intervento, a cui avevo già accennato, è quello più propriamente medico-scientifico, cioè il potenziamento degli strumenti e il fatto di rendere accessibili le nuove terapie superando le diseguaglianze, necessità di aggiornare le tecnologie, il cosiddetto parco macchine degli ospedali che spesso è obsoleto ed insufficiente per le necessità. dell'assistenza territoriale. Forse non tutti sanno che da decenni in oncologia la parola d'ordine è «decentrare», cioè assistere le persone il più possibile vicino ai loro ambienti di vita, il più possibile nelle famiglie. Questo aspetto è stato sottolineato da molti.

è pertanto impossibile farne funzionare una parte se tutto il sistema non viene reso in grado di operare bene Dovendo provvedere a una ricostruzione del nostro sistema sanitario, risollevandolo dal disagio in cui si trova adesso, dovremmo pertanto pensare anche ai tagli che ci sono stati negli ultimi anni.

Signor Presidente, gentili colleghi, il prezzo che abbiamo pagato fino ad oggi in questa pandemia e che continueremo a pagare in termini di vite umane fino al giorno della raggiunta immunità di gregge è solo un assaggio di quello che ci aspetta. Il giorno in cui ne saremo fuori faremo i conti con la peggiore delle ondate, quella che porta il nome e la sofferenza delle centinaia di migliaia di pazienti che hanno avuto in sorte di contrarre malattie gravi, potenzialmente letali e invalidanti come e più del Covid, alla vigilia o nel corso di questo anno e mezzo di pandemia. Si tratta di malati che non hanno avuto più reparti ospedalieri in cui ricoverarsi, o che hanno visto diradarsi, fino a scomparire, visite specialistiche ed esami che avrebbero potuto diagnosticare tumori prima che le loro metastasi li rendessero non più aggredibili. È noto, infatti, che la diagnosi e il trattamento precoce del tumore primitivo migliorano notevolmente la prognosi *quoad vitam* talvolta radicalmente. Numeri alla mano,

con un ritardo di diagnosi i cui effetti nefasti si vedranno nel tempo. Lo *screening*, infatti, rappresenta un momento fondamentale in oncologia poiché l'anticipazione diagnostica è ancora oggi uno dei principali fattori che migliora la prognosi e una delle armi, specie in alcune tipologie di tumore come quelli della mammella, del colon e della cervice uterina. Purtroppo ancora oggi la maggior parte dei casi di tumore viene identificata solo quando compaiono i sintomi meritevoli di approfondimento diagnostico, di solito in ambito ospedaliero. Nel periodo del *lockdown* l'accesso all'ospedale e alle attività diagnostiche si è drasticamente ridotto non solo per motivi oggettivi, quali la difficoltà nella differenziazione dei percorsi, la scarsità di risorse umane e le carenze tecnologiche, ma anche per la paura dei pazienti a recarsi presso le strutture ospedaliere. Le Regioni, in modo comunque eterogeneo, hanno cercato di garantire il percorso oncologico al fine di assicurare, per quanto possibile, i trattamenti chemioterapici, le terapie chirurgiche e i trattamenti di radioterapia. In linea generale, sono state implementate tutta una serie di attività emergenziali, quindi con caratteristiche di sperimentazione sul campo, che hanno comunque consentito di mantenere il contatto con il paziente oncologico. Solo alcune iniziative si sono avvalse dell'utilizzo della telemedicina: si pensi alla gestione di alcune visite di *follow-up* a livello territoriale o alla domiciliazione di alcune terapie chemioterapiche. iniziative sono servite a cercare di mantenere il rapporto tra medico e paziente, ma allo stesso tempo hanno messo in moto una profonda accelerazione di un processo che ormai da qualche anno iniziava ad avere un'evidenza, ossia cominciare a ripensare l'oncologia nell'ottica di una più forte integrazione tra ospedale

al quale riferirsi ed è anche uno degli elementi fondamentali con i quali si stanno declinando le reti per patologia all'interno della rete oncologica. La rete oncologica non può basarsi, infatti, solo sul coordinamento tecnico-professionale fatto da esperti o da figure competenti, ma deve essere una vera e propria struttura organizzativa con alla guida figure chiave da un punto di vista gestionale che alimentino e gestiscano tutti i diversi livelli organizzativi interaziendali. Si tratta di una dimensione meta-aziendale che consente di poter unire, all'interno di una rete per patologia, le modalità con cui tutti i protagonisti sono chiamati a interagire, avendo un unico riferimento concettuale ed organizzativo. Tempi di reazione e *governance* dei rapporti tra territori e strutture ospedaliere dipendono molto dal livello di strutturazione che ciascuna Regione riesce a consolidare per la propria rete oncologica che la pandemia ha messo a dura prova. La seconda fase della pandemia da Covid-19 non ci ha colto però così impreparati, e pertanto, nonostante l'incremento consistente dei ricoveri Covid, si è osservata una graduale ripresa delle attività cliniche fondamentali non-Covid. Da questa esperienza dobbiamo trarre molti spunti per dare una forte spinta all'innovazione organizzativa all'interno dei nostri sistemi sanitari. Le modalità alternative, soprattutto per quanto riguarda gli accessi ambulatoriali, hanno costituito un terreno di prova importante per tutto quello che è ormai riconducibile all'*e-Healt*, e quindi non soltanto le televisite e il teleconsulto, ma anche la possibilità di monitorare i pazienti al proprio domicilio. Sappiamo però tutti che la telemedicina è un po' come la didattica a distanza: non può essere sostitutiva dell'assistenza, ma integrativa. L'esigenza di un nuovo Piano oncologico nazionale, fermo al 2016, è adesso quanto mai attuale in quanto strumento per disegnare le linee guida nazionali dallo *screening* fino alle cure palliative. Quando infatti si parla di oncologia, non si possono trascurare tutti i *setting* assistenziali correlati; non possiamo parlare solo di quello ospedaliero o di quello domiciliare, soprattutto se vogliamo traguardare il tutto attraverso il concetto di rete. Il nuovo Piano nazionale dovrà incidere sui temi della genomica, delle mutazioni spontanee e sull'anticipazione degli *screening* per familiarità, garantendo quel tanto auspicato salto di qualità dell'oncologia nazionale. È necessaria una reazione a trecentosessanta gradi immediata, e oggi noi qui riuniti siamo a testimonianza del nostro impegno per garantire ai pazienti oncologici i migliori *standard* di diagnosi e cure, nonostante si sia nella terza ondata pandemica che continua ad assorbire risorse in un modo straordinario. I tristi bollettini giornalieri dei decessi e contagi da Covid-19 hanno occupato la scena dei *mass media*, ma non dobbiamo dimenticare il numero ben più alto delle persone che muoiono tutti i giorni per malattie croniche, per tumore e per patologie cardiovascolari. Il secondo elemento è l'assistenza territoriale in continuità con l'ospedale. Le USCA saranno la struttura portante della continuità assistenziale; all'interno di questi gruppi, una volta che finirà la pandemia, ci dovranno essere anche gli specialisti e tra questi gli oncologi territoriali, oltre che gli psicologi e i terapisti del dolore. Se infatti vogliamo parlare di assistenza domiciliare oncologica, non può essere solamente di tipo infermieristico. Un discorso a parte meritano gli *screening*. Lo *screening* oncologico è un servizio che viene offerto gratuitamente ai cittadini italiani, però questa risorsa è utilizzata - quando va bene e, soprattutto, a certe latitudini - al massimo dal 25 al 30 per cento delle persone alle quali è rivolto, il che significa che abbiamo circa il 70 per cento di strategia preventiva che ha un costo, ma è sottoutilizzata. Il professor Sileri ci insegna quale differenza ci sia tra un polipo del colon in primo stadio e una situazione invece avanzata di un cancro del colon e in questo lo *screening* rappresenta l'arma vincente. Dobbiamo quindi tornare indietro per rimettere l'attenzione sull'utilità dei Dipartimenti di prevenzione, non solo in campo vaccinale. Dal punto di vista dell'organizzazione del sistema sanitario, nonché dal punto di vista delle opportunità che può offrire al sistema di *welfare* nel suo complesso, la pandemia deve darci degli spunti di riflessione circa lo sviluppo di un nuovo rapporto tra ospedale e territorio, se consente di elaborare e seguire dei dei percorsi diagnostico-terapeutici appropriati. La creazione di percorsi diagnostico-terapeutici definiti consentirebbe una razionalizzazione della spesa e una migliore gestione del paziente all'interno del territorio dove la rete oncologica opera. Un cenno, infine, vorrei farlo sul sistema della mobilità extra-Regione. Il problema presto esploderà, perché la mobilità nel 2020 si è quasi azzerata e nel 2021 continuerà a essere molto bassa. Come faranno allora le Regioni che prima mandavano tutti i pazienti fuori ad assisterli in maniera corretta? Bisognerà capire se queste Regioni e le loro strutture sanitarie saranno o meno in grado di fornire questo tipo di assistenza e, ove non lo fossero, bisognerà investire da subito controllando e monitorando, verificando tutto, affinché si possa garantire una gestione corretta del paziente oncologico. Per concludere, ritengo che la pandemia sul piano organizzativo possa considerarsi come un punto di svolta e di accelerazione di alcune attività su cui si stava già lavorando, perché il mondo non è più lo stesso. È quindi necessaria la creazione e l'ottimizzazione delle reti oncologiche regionali come strumento per la corretta presa in carico multidisciplinare del paziente, l'individuazione di percorsi diagnostico-terapeutici strutturati che garantiscano il funzionamento della rete e la gestione del paziente oncologico e l'investimento negli strumenti della telemedicina, vista come il completamento utile e necessario alla gestione del paziente, con particolare riferimento al *follow-up.*

Signor Presidente, signori Sottosegretari, onorevoli colleghe senatrici e colleghi senatori,

Signor Presidente, signori Sottosegretari, onorevoli colleghe senatrici e colleghi senatori, la grave la grave pandemia da Covid-19 sta mettendo a dura prova la tenuta del Servizio sanitario nazionale, provocando, oltre a un considerevole eccesso di mortalità, un progressivo aumento del numero dei malati oncologici, costretti a ritardare controlli e a rimandare le proprie cure. La prevenzione terziaria, quella mirata all'anticipazione diagnostica della ripresa di malattia, non è procrastinabile nei pazienti oncologici, perché la mancata tempestività della diagnosi di ripresa comporta minori possibilità di guarigione, con il conseguente aumento del numero di anni di vita persi. Oggi oltre il 50 per cento dei malati oncologici guarisce definitivamente e un'altra parte consistente cronicizza la propria malattia per effetto delle cure, conseguendo traguardi di aspettativa di vita e di lunga sopravvivenza pressoché pari a quelli in assenza di malattia. Oltre alla prevenzione terziaria, anche la prevenzione secondaria, ovvero quella rivolta agli *screening* nella popolazione sana, risente fortemente delle attuali condizioni di emergenza sanitaria e ciò non dovrebbe accadere, perché è risaputo che un ritardo nella diagnosi di un tumore comporta interventi terapeutici più complessi e aggressivi, con ulteriore detrimento delle condizioni psicofisiche dei pazienti e aumento dei costi sanitari. A rendere più gravi queste situazioni, come già detto, si aggiungono spesso condizioni di disagio economico e di non meno importante disagio psichico, che peggiorano la qualità di vita dei pazienti oncologici, compromettendo gli sforzi sociali e individuali tesi al superamento della malattia. Non vi è dubbio che l'attuale malattia stia mettendo a dura prova i risultati conseguiti negli anni passati nella lotta al cancro attraverso gli interventi di prevenzione primaria e secondaria messi in atto dal nostro sistema sanitario. Il miglioramento del nostro servizio sanitario passa soprattutto dal potenziamento della medicina territoriale, a partire dalle cure domiciliari, che devono divenire primo e appropriato luogo di cura per ridurre accessi impropri alle strutture ospedaliere, avvalendosi dei vantaggi e dei benefici offerti dalla telemedicina e dalle altre tecniche di sanità digitale. In tale contesto non possono essere trascurate prevenzione e cura delle malattie oncologiche, per le quali si rendono indifferibili l'aggiornamento del Piano oncologico nazionale e il potenziamento e l'interconnessione delle reti oncologiche regionali. Le reti sono strumenti indispensabili per la presa in carico globale dei pazienti oncologici; favoriscono appropriatezza e qualità delle cure ed economie di scala del sistema sanitario nazionale e aumentano anche la fiducia e l'adesione dei malati al sistema. Per un efficace e adeguato funzionamento delle reti è fondamentale la conoscenza dei dati relativi alle malattie oncologiche trasmesse dai registri tumori. Pertanto, come ha giustamente osservato in apertura il sottosegretario Sileri, occorre dare esito alla pubblicazione del regolamento esecutivo per l'attuazione della legge del 22 marzo 2019, entrata in vigore il 20 aprile 2019, relativa appunto all'istituzione della rete nazionale dei registri tumori, per la quale peraltro è già stato previsto uno stanziamento di un milione di euro dalla legge di bilancio del 2020. Accessibilità alle reti e organizzazione delle reti sono due pilastri sui quali si regge un'efficace attività sanitaria di contrasto alle malattie oncologiche, unitamente alla ricerca, che costituisce un terzo importante pilastro. La ricerca in campo oncologico ha compiuto numerosi e importanti progressi, conseguendo obiettivi di cura impensabili fino a pochi anni addietro attraverso le scienze omiche. Gli studi di genomica, proteomica e metabolomica hanno consentito di confezionare terapie personalizzate sui singoli pazienti, portando a livello intracellulare le possibilità di intervenire terapeuticamente e di correggere gli errori alla base della nascita e della crescita tumorale delle cellule. Per tale motivo si ritiene indispensabile anche l'attuazione del Piano per l'innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche medicina personalizzata, sancito nell'intesa Stato-Regioni il 26 ottobre 2017, al fine di garantire ampio accesso alla medicina di precisione e di promuovere investimenti finalizzati alla formazione di personale specializzato e alla creazione di strutture adeguate. L'aggiornamento del Piano oncologico nazionale non può essere disgiunto dall'ampliamento dell'offerta di terapia del dolore e di cure palliative, come già richiesto da mozioni presentate dalla Commissione sanità, impegnando il nostro Governo. Ai fini di un efficace trattamento del dolore e della sofferenza, anche l'offerta di cure palliative deve avvenire prioritariamente, ove possibile, a domicilio del paziente, nella sua casa, nel suo ambiente quotidiano di vita, con il sostegno psicologico e spirituale anche alla famiglia, sulla quale quasi sempre grava il maggiore peso assistenziale, proprio nel momento di maggiore fragilità psichica. In ultimo, non può essere sottaciuto che nel Piano oncologico nazionale sarà necessario rivedere l'assetto delle reti oncologiche regionali, affinché siano ridotte e annullate le differenze attualmente esistenti tra le varie Regioni e Province autonome, con il superamento di centri e comitati di controllo regionali, spesso causa di inopportuni ritardi, e siano stabilite quindi modalità di accesso unitarie e omogenee in tutto il territorio nazionale contemporaneamente, ivi compresa la disponibilità e la fruibilità dei farmaci. Disomogeneità regionali che si eviterebbero con il ritorno alle competenze esclusive dello Stato in tutti gli interventi in materia di sanità. L'Italia ha bisogno di questo nuovo Piano oncologico nazionale, perché quello attuale è scaduto da anni e risulta superato peraltro dai progressi della scienza e della tecnica. Pertanto riteniamo che sia oggi necessario non farci trovare impreparati a questa sfida e che sia doveroso prevedere un impegno per il Governo finalizzato all'adozione del nuovo Piano oncologico nazionale, coordinato con il piano oncologico europeo. Come MoVimento 5 Stelle crediamo che l'equità di un sistema sanitario si evinca dal trattamento e dall'attenzione che riserva ai soggetti più fragili.

del voto in dissenso per denunciare un fatto grave, che mi sembra però importante. «Svegliati amore mio» è una *fiction* andata in onda sulle reti Mediaset, quale si racconta la tragedia di chi vive certe situazioni in cui si deve scegliere tra il diritto al lavoro e il diritto alla salute, e anche il diritto a non dover morire proprio di tumore. Su questa *fiction* televisiva un lavoratore ha espresso un'opinione e ha postato sulla propria pagina Facebook l'invito a guardarla, commentando proprio il diritto in questione,

Ecco, questo lavoratore è stato licenziato per avere condiviso sulla propria pagina Facebook un'opinione rispetto al dover scegliere, in queste città, tra il diritto al lavoro e quello alla salute. Era importante che, in un'occasione del genere, si sottolineasse la gravità assoluta di questo fatto. Ora, se mi perdonerete

la migliore, anche perché non mancano occasioni parlamentari per poter far presente un argomento che è sicuramente importante.

Signor Presidente, annuncio che stiamo definendo un ordine del giorno unitario, quindi sono pronta a ritirare la mozione non appena

Colleghi, per cortesia, consentiamo alla senatrice di svolgere il suo intervento.

poiché attiene alle priorità vaccinali, di cui tanto abbiamo discusso in questo anno e in questi ultimi giorni. Decidere chi vaccinare prima e chi dopo, in mancanza di dosi sufficienti per l'intera popolazione,

La mozione chiede anzitutto di implementare il piano vaccinale del commissario straordinario Figliuolo, di eliminare le differenze tra le Regioni, a cui assistiamo, purtroppo, ancora in questa fase,

Comunque sia, vi prego di seguire con più attenzione, fermo restando che non c'è tutto questo disturbo, siamo in pochi.

implica scelte etiche che questo Parlamento ha tutta la responsabilità di prendere.

in cui si afferma che, in caso di profilassi internazionale, le cure e gli interventi per le epidemie sono esclusivamente in capo allo Stato.

è più pesante si perde il tracciamento e pensiamo di doverlo riprendere, soprattutto per le famiglie con figli che stanno ricominciando ad andare a scuola. L'altra questione riguarda i dati: preghiamo il Governo di fare una riflessione attenta

chiudere repentinamente zone anche circoscritte in cui riparte l'epidemia e di riaprire quando le condizioni migliorano, potremmo anche evitare di chiudere intere Regioni. Dati aggiornati e tracciamento devono quindi accompagnare la campagna vaccinale.

Abbiamo appena approvato un ordine del giorno con il quale vogliamo difendere i malati non Covid da una sorta di ipertrofia che attraversa il Paese, per cui tutto viene letto con gli occhiali da Covid,

tende a sottolineare tre cose, che vorrei risultassero chiare. La prima è che oggi il vaccino, proprio perché rappresenta una sorta di misura salvavita, diventa parte integrante del diritto alla salute, che non soltanto è contemplato dalla nostra Costituzione, ma è anche previsto tra i diritti universali dell'uomo.

chiusi in casa dalla didattica a distanza o a coloro che stanno aspettando, con grande attenzione, che riapra tutto il grande mondo della produzione; percepiamo questo tema soprattutto sotto il profilo della distribuzione, è evidente però che c'è tutta la produzione. Penso poi anche al mondo del turismo, eccetera. Tutto dipende dunque dal diritto alla salute, che può essere garantito attraverso il diritto alla vaccinazione.

quindi un diritto cerniera tra quelli individuali e quelli sociali e ci permette di ripensare l'intera gamma dei diritti, in una logica solidaristica molto più ampia e molto più profonda. Se tutto questo è vero, allora è fondamentale che in tempo di pandemia si possa sospendere - non abolire, ma sospendere - il brevetto della vaccinazione. A proposito dunque della brevettabilità dei prodotti, che molto spesso guarda anche

il diritto alla proprietà intellettuale, che va custodito, protetto e tutelato, possa però essere sospeso nel momento in cui diventa una *conditio sine qua non* per il diritto alla vita di molte persone.

nell'ordine del giorno unitario. Se esso conterrà questi punti, posso ritirare tranquillamente la mia mozione e farla convergere in un obiettivo condiviso con tutta l'Assemblea. Signor Presidente, illustro la mozione presentata dal MoVimento 5 Stelle e a prima firma del senatore Romano. Stiamo vivendo un nuovo capitolo di questa pandemia: il primo anno ci siamo concentrati a ridurre il contagio, per ridurre i ricoveri e quindi il numero di decessi, e adesso l'obiettivo dev'essere somministrare quanti più vaccini possibile, per ripartire. Per la prima volta abbiamo un vaccino che è stato acquistato con una gara d'appalto unica a livello europeo, proprio per garantire un accesso equo, diffuso e ripartito esclusivamente in base al numero dei cittadini di ogni Paese.

In questo momento storico, infatti, il nazionalismo certamente non aiuta. Anche l'Organizzazione mondiale della sanità ha chiesto un'equa distribuzione dei vaccini e Amnesty international ha denunciato atteggiamenti opportunistici di diversi Paesi nell'acquisto dei vaccini. Mai come in questo momento nessuno si salva da solo; in un momento in cui le disuguaglianze sono aumentate, se aumentano anche quelle nella somministrazione dei vaccini, mettiamo a rischio la ripartenza di alcuni Paesi e possiamo creare divari che non saranno più recuperabili in termini sia di vite perse sia di PIL. Bisogna poi fare presto, perché

infettare i soggetti guariti, evadendo in qualche modo la risposta immunitaria da Covid. Ecco perché serve fare presto e non basta esclusivamente bloccare l'*export* dei vaccini, ma bisogna aumentarne la produzione. produzione. Succede oggi che uno Stato che cofinanzia un brevetto non ha alcuna voce in capitolo né sul costo, né sulla vendita, né sulla distribuzione del prodotto. Ecco perché in questo momento storico, in cui il mondo è cambiato, dobbiamo ribaltare anche tale prospettiva e garantire ai Paesi uno spazio decisionale *(Applausi)* per coprire il fabbisogno vaccinale.

utilizzando anche lo strumento della licenza obbligatoria, arma negoziale importante con le case farmaceutiche. Molti Stati lo hanno già fatto; la Germania, ad esempio, ha rafforzato lo strumento della licenza obbligatoria.

in testa. Alla Camera dei deputati è già stata approvata una mozione che spinge l'Europa ad approvare tale normativa e con questo testo chiediamo un impegno anche al Senato.

stiamo parlando ancora una volta del tema dei vaccini. Giustamente, come hanno ricordato prima i colleghi, in questi giorni - e

Come dicevo, le criticità che purtroppo sono emerse in questa pandemia le riscontriamo tutte in questo momento. Il commissario Figliuolo, come sapete, ha girato per tutti i punti vaccinali del territorio nazionale e ha trovato anche delle eccellenze,

ha detto lui, come avete visto anche nei TG. Ciò significa che si può fare, nel senso che organizzare bene le strutture e il personale è possibile. Credo che anche da questo punto di vista le *best practice* vadano copiate,

trovato vaccini per combattere il Covid, però le criticità ci sono; ritengo tuttavia che anche oggi stiamo dando un buon segnale per trovare tutti insieme modalità nuove e spunti ulteriori da dare al nostro Governo *(Applausi)*.

parliamo finalmente del piano vaccinale, argomento su cui questo Parlamento anestetizzato è stato sin qui tenuto ai margini. Tuttavia, per parlare seriamente di tale argomento, che necessita indiscutibilmente di un approccio scientifico, occorre preliminarmente affrontare il tema della trasparenza dei dati scientifici e della terzietà e imparzialità rispetto al potere politico degli organismi scientifici che tali dati sono chiamati a interpretare. Si è recentemente scoperto, infatti, che il piano pandemico, che avrebbe dovuto proteggere il Paese dalla diffusione del Covid e che avrebbe potuto evitare moltissime perdite di nostri cari, non era mai stato aggiornato: giaceva semplicemente in qualche cassetto da decenni. questa vicenda sta facendo emergere una clamorosa assenza di terzietà ed autorevolezza da parte dei vertici delle più importanti organizzazioni medico-scientifiche, che dovrebbero fornire dati e informazioni a prescindere dal fatto che ciò piaccia o dispiaccia al potere politico. Se è infatti appreso, signor sottosegretario Sileri, dalla pubblicazione di alcune intercettazioni tra il vice presidente dell'Organizzazione mondiale della sanità, già direttore generale del Ministero della salute, Ranieri Guerra, e il Presidente dell'Istituto superiore di sanità, nonché attuale membro del CTS, che il *report* dei ricercatori dell'ufficio regionale dell'OMS con sede a Venezia, coordinati dal professor Zambon, era stato occultato per non dispiacere alla sensibilità politica del ministro Speranza, con il coinvolgimento diretto del capo di Gabinetto di tale Ministero e, con ogni probabilità, anche del ministro Speranza. Le intercettazioni sono agghiaccianti e inequivocabili: i vertici dei due organismi scientifici chiamano i ricercatori "gli scemi di Venezia", i "somarelli di Venezia" e si rassicurano l'un l'altro di essersi profusi in scuse profonde con il Ministro per un *report* che, dicendo la verità, avrebbe gettato discredito sul suo operato.

sottosegretario Sileri, comprenderà che su questa vicenda si gioca la credibilità delle istituzioni scientifiche su cui il suo Ministero basa le proprie azioni. Sembra infatti evidente che il suo Ministero abbia influenzato importantissime risultanze scientifiche che avrebbero potuto compromettere l'operato del Ministro e tutto questo grazie alla lottizzazione dei ruoli apicali in tali organizzazioni e all'assenza di garanzie di terzietà tra politica e mondo scientifico-sanitario. Su questo, il ministro Speranza sta evitando di rispondere anche a interrogazioni che sono state presentate in quest'Aula, ma tale mancanza di trasparenza non vi è nuova: c'è già stato lo scandalo per le secretazioni dei verbali del CTS, sbloccati solo grazie ad un'ordinanza del TAR del Lazio; e vogliamo parlare della trasparenza nelle regole di approvvigionamento dei vaccini e delle norme contrattuali che ne regolano l'acquisto? Questi contratti sono avvolti dal segreto, avvantaggiando enormemente i profitti dei produttori di vaccini. La stessa assoluta mancanza di trasparenza ha contraddistinto anche il caso AstraZeneca, in cui gli organismi scientifici e il Governo hanno negato fino all'ultimo il nesso con le trombosi, salvo poi arrendersi all'evidenza e limitarne l'uso a determinate determinate fasce d'età. Alla luce di tale opacità delle informazioni scientifiche e di una narrazione da parte di alcuni vertici delle organizzazioni scientifiche preposte alla salute che tiene conto della sensibilità governativa, risulta difficile giudicare compiutamente alcune delle azioni del Governo. È però lecito dubitare delle eccessive delle eccessive restrizioni delle ultime settimane e anche che venga sottorappresentato il calo stagionale che il virus sta avendo a prescindere dalle restrizioni e dalla campagna vaccinale. Qualcosa, però, si può dire con certezza. però, si può dire con certezza. Non ci sono certezze sulla capacità dei vaccini di interrompere il contagio, ma solo di evitare le conseguenze peggiori sui vaccinati e, poiché è certo che l'età media dei morti per Covid è di ottantun anni, risulta evidente che si sarebbe dovuto procedere vaccinare prima le classi di età maggiore e i più fragili e non a seconda delle categorie lavorative, quindi non solo quanto al reperimento è risultato fallimentare questo piano, ma si sono vaccinate le persone sbagliate, con il risultato che siamo al secondo posto per morti.

nei confronti del vice presidente dell'OMS, voterà contro le mozioni presentate e chiede la costituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare sulla gestione della pandemia. *(Applausi)*. PRESIDENTE. Non l'ho interrotta, ma la prego, la prossima volta, di non usare termini sconvenienti.

su cui si gioca il concetto di sovranità. Questo significa che la guerra per gli approvvigionamenti e per le dosi del siero è in atto. Noi, naturalmente, confidiamo nel presidente Draghi e nella struttura commissariale, impegnata ad ottenere 10 milioni di dosi aggiuntive rispetto al previsto. Ma è di oggi la notizia dell'arrivo di 45 milioni di dosi entro giugno: così la campagna vaccinale sarebbe salva. Confidiamo intanto nella produzione dei vaccini italiani (Takis, Reithera) prodotti in collaborazione con lo Spallanzani di Roma, che ha completato già la prima fase. L'obiettivo è produrre un vaccino monodose, di cui a settembre potrebbero essere disponibili ben 100 milioni di dosi. Quindi voglio essere ottimista e fiduciosa: tutte le epidemie hanno un inizio e una fine. Ma la domanda che noi tutti ci poniamo è: quando, grazie ai vaccini, l'Italia potrà ripartire? È più realistico puntare su un abbassamento della letalità oppure sperare nell'immunità di gregge? L'immunità si raggiungerà soltanto quando si riuscirà a bloccare la circolazione del virus. Se avessimo un vaccino efficace al cento per cento contro il contagio e la certezza di una copertura duratura, il risultato potremmo averlo vaccinando il 70 per cento della popolazione. Ma i vaccini Pfizer e Moderna hanno un'efficacia del 97 per cento e Astrazeneca del 60-80 per cento. Adesso è arrivato anche Johnson & Johnson, che può essere somministrato dai diciotto anni in su, con efficacia fino al 77 ma per ora - è notizia di oggi - è stato sospeso negli Stati Uniti per gli effetti sulla coagulazione del sangue. L'immunità di gregge potremmo raggiungerla soltanto vaccinando il 97 per cento della popolazione. Ma se consideriamo che ci sono tante persone contrarie al vaccino e che proprio non intendono vaccinarsi, e che non sappiamo ancora quanto durerà l'immunità, la famosa immunità di gregge sarà per ora un miraggio.

Dopodiché la letalità si abbasserà notevolmente e diventerà simile a quella dell'influenza. Ma tutto ciò sarà possibile solo se Pfizer, Moderna e Astrazeneca rispetteranno i termini di consegna dei vaccini, le diffidenze su Astrazeneca si placheranno e se il piano del commissario Figliuolo procederà rapidamente raggiungendo le 300.000 dosi entro fine aprile e le 500.000 inclusi i richiami. Certo dobbiamo avere fiducia, ma è già polemica sulle isole, che vorrebbero presto diventare Covid *free* insieme alle piccole isole. La richiesta del presidente Solinas e del presidente Musumeci di dare priorità al piano vaccinale in Sardegna e Sicilia per rilanciare il turismo, e raccolta anche dal ministro Garavaglia, ha fatto infuriare il presidente Bonaccini. Per me è una richiesta lecita, viste le condizioni di svantaggio che si avvertono quando si vive in un'isola, che ci penalizzano soprattutto sul piano infrastrutturale. senza polemiche, intanto trovo giusto che ci si concentri sulle vaccinazioni, affinché avvengano nel più breve tempo possibile e si lavori perché in tutta Europa si possa avere il certificato Green digitale. Si pensi, soprattutto, a sostenere la ricerca nel campo degli anticorpi monoclonali. mi permetta, signor Presidente, di fare tanti auguri di buon lavoro alla dottoressa Maria Chiara Carrozza, che sarà la prima donna alla guida del CNR che finalmente, dopo aver subito numerosi tagli, tornerà a svolgere al meglio le sue funzioni organizzative, e scientifiche. In questo particolare momento abbiamo bisogno di potenziare e finanziare la ricerca. Mi riferisco proprio agli anticorpi monoclonali, il cui utilizzo può essere di grande aiuto. L'obiettivo sarà proprio quello di verificare se potranno rappresentare una reale terapia per la prevenzione e la progressione della malattia stessa. Ricordo che gli anticorpi monoclonali sono utilizzati principalmente in clinica e...

la pandemia ha veramente posto tutti noi in una situazione di estrema difficoltà, non solo in Italia, ma nel mondo intero.

Il Coronavirus ha messo in evidenza molte debolezze della nostra struttura sanitaria. Purtroppo è successo che nella fase iniziale, al di là delle informazioni che venivano date, le persone si recassero, come erano solite fare, in ambito ospedaliero. Questa situazione è stata di estrema gravità perché l'afflusso eccessivo di pazienti in ospedale ha determinato un'ulteriore diffusione della malattia. Come sappiamo, l'ospedale è un centro di alta specializzazione, dove si devono curare necessariamente i pazienti che hanno specifiche necessità di essere assistiti. Tuttavia, la presenza di molti pazienti all'interno dell'ospedale

avevo presentato un disegno di legge, che è incardinato in Commissione sanità, riguardante la figura dell'infermiere di famiglia. Lei sa benissimo, e lo sappiamo tutti, quanto sia importante il ruolo dell'infermiere di famiglia o di comunità.

essere effettuate sui pazienti a rischio e sul personale sanitario; mi corre l'obbligo di dire che tutti i sanitari e tutti quelli che gravano nell'ambito ospedaliero devono necessariamente essere

ringrazio tutti i colleghi che hanno lavorato alla stesura di questo ordine del giorno e ringrazio il Governo per aver partecipato. L'invito, sottosegretario Sileri, è quello di

Lo dico perché reputo intollerabile che si possa dare rappresentanza politica o istituzionale a chi vuole scavalcare la fila

Prima si è immaginato di utilizzare la categoria «altri», che era stata individuata in Parlamento e dal Governo per dare mandato alle Regioni per stabilire quali potessero essere le tipicità su cui intervenire, oltre alle professioni sanitarie, che reputavamo fossero quelle che necessitavano prima di tutte di essere vaccinate. è così utilizzata quella categoria «altri» per privilegiare alcune professioni. Strano, ad esempio, che non siano rientrate mai tra le professioni da vaccinare prioritariamente le commesse e i commessi, che nemmeno in pieno *lockdown*, quello più spinto, hanno mai smesso di lavorare. C'è però stato questo tentativo e credo che

zone franche in cui anticipare la vaccinazione e, anche in quel caso, utilizzare lo strumento per scavalcare la fila, non comprendendo che l'unico modo per rendere un luogo Covid-*free* è l'immunità di massa. Infatti, anche se vaccinati si è contagiosi, signor Sottosegretario.

Io credo che l'unico elemento cui dobbiamo fare riferimento per stabilire le priorità siano i dati oggettivi, purtroppo, dei deceduti in questi tredici mesi di pandemia.

Credo, quindi, che l'unico criterio oggettivo da utilizzare sia la vaccinazione prioritaria delle persone incluse in fasce d'età particolari e in condizioni particolari di fragilità e di disabilità. questo debba essere l'unico criterio che ci dobbiamo dare per proseguire nella vaccinazione. Il secondo obiettivo da centrare è, poi, l'immunità di gregge, proseguendo sempre per fasce d'età, come è stato ribadito anche oggi dal ministro Gelmini e noi condividiamo pienamente. Naturalmente, per raggiungere l'immunità di gregge, è possibile utilizzare degli strumenti.

Dobbiamo evitare il limite di chi ogni volta programma gli strumenti di cui si deve dotare nel momento stesso in cui ne ha bisogno; vanno già da ora stabilite le modalità e le norme per la *privacy* che dovremo assolutamente rispettare. rispettare. Lo strumento del passaporto inoltre sarà un incentivo alla vaccinazione e la speranza è che per raggiungere l'immunità di gregge non si debba mai arrivare all'obbligo vaccinale, ma, se l'obiettivo è quello,

Se questo è vero, se noi sommiamo alla campagna vaccinale l'estate alle porte (abbiamo già visto che l'estate passata è stata una stagione che ha conosciuto una drastica riduzione dei contagi), se mettiamo insieme queste due azioni, noi possiamo dire che le prossime saranno le giornate della ripartenza per questo Paese.

e la calendarizzazione con date certe ci consentirà anche di evitare brutte figure e dannose, come la riapertura promessa per la stagione sciistica e mai mantenuta, con costi enormi di cui le imprese si sono dovute caricare. Accanto a questo naturalmente pensiamo che bisogna continuare con le azioni a sostegno delle imprese e dei lavoratori con il decreto-legge sostegni 2 e con le misure che saranno necessarie. Questi sono gli unici strumenti per fermare le proteste, che sono legittime se pacifiche, vista la condizione economica di questo Paese. Già oggi, Sottosegretario, si può programmare la stagione turistica: possiamo dire che si andrà in vacanza in Italia, possiamo dire agli italiani che possono chiamare le agenzie di viaggio e prenotare la vacanza, perché questa è una condizione oggettiva a cui si potrà giungere.

servono 30 miliardi di investimento sulla sanità per potere garantire anche chi oggi non può permettersi cure, perché la nostra struttura sanitaria è fisiologicamente oberata

che investire in sanità sia assolutamente indispensabile così come investire nella sensibilizzazione per la campagna vaccinale. La politica non deve mettere "il becco" sulla valutazione dei vaccini. La valutazione della bontà scientifica di un vaccino spetta all'EMA e all'Aifa in Italia, non ai Paesi

Gli Stati Uniti decidono di interrompere, ma gli Stati Uniti hanno 300 milioni di dosi messe a disposizione da Moderna e Pfizer. Se in Italia e in Europa si sospende Johnson & Johnson e AstraZeneca senza alcun motivo scientifico, si interrompe la vaccinazione e si crea un enorme danno al Paese. necessaria un'azione che riguardi una campagna di sensibilizzazione forte, da accompagnare alle misure

dall'altro dobbiamo a tutte le famiglie vittime del Covid la verità sugli errori commessi e sulle responsabilità per una situazione che, da certi punti di vista, ci è anche un po' sfuggita di mano.

in questo momento storico. Abbiamo sempre detto, e lo ha sempre ribadito il nostro presidente Giorgia Meloni, che avremmo avuto questo atteggiamento nei confronti dell'attività di Governo,

campagna vaccinale e cioè, sostanzialmente, "all'ultima spiaggia", ovvero all'ultima possibilità di recuperare il tanto tempo perso e i tanti errori fatti.

Grazie, dalla nostra classe medica e da tutto il personale impegnato nell'emergenza Covid. Li abbiamo pagati, soprattutto, con una quantità enorme di crisi industriali, di posti di lavoro persi

abbiamo detto mille volte in Commissione, che quello che è accaduto, dalla dichiarazione dello stato d'emergenza ad oggi, debba essere affrontato e analizzato seriamente e lucidamente da una Commissione parlamentare di inchiesta. È ovvio che, rispetto a quello che sta accadendo, non possiamo fare da semplici spettatori distratti, o peggio interessatamente disinteressati: scusate il conflitto apparente di termini. Dobbiamo convincerci della

evidentemente tutte le strutture e accelerando tutti i processi di invecchiamento di tale provvedimento. Il microfono continua a lampeggiare, Presidente, è una sorta di intimidazione

La parte essenziale è che noi, con la stessa onestà con cui dobbiamo ammettere che tanti errori sono stati compiuti, analogamente dobbiamo riconoscere, colleghi, che la parte che manca in questa enorme azione di campagna di vaccinazione è il vaccino. Abbiamo oggi, dove meglio e dove peggio, le Regioni che hanno risposto con i propri piani vaccinali e si sono attrezzate ad erogare e somministrare

Acclarata la circostanza non del tutto irrilevante che abbiamo preparato la mitragliatrice, come ho detto al generale Figliuolo, ma non abbiamo predisposto le munizioni, per cui ci siamo messi dentro un accordo - che andremo a valutare quando e se

di fronte ad una grave circostanza: dobbiamo immediatamente attivare ogni possibile canale per aumentare la disponibilità dei vaccini da trasferire alle Regioni, che sono pronte a somministrarli. Continuiamo a intrattenerci, sembra che ne abbiamo la volontà, con una sorta di azione di distrazione di massa; continuiamo infatti ad impegnarci su chi deve vaccinare, su chi deve vaccinare, dove e come dobbiamo vaccinare, sullo scudo penale da riconoscere ai vaccinatori, se devono vaccinare i farmacisti o i dentisti, e su tutta una serie di discussioni, che però risultano ampiamente sterili nel momento in cui noi non diamo la disponibilità dei vaccini. Mi rivolgo al rappresentante del Governo, consapevole più di me che un collo di bottiglia che sta strozzando l'intera campagna vaccinale. Il primo passaggio importante di questo ordine del giorno è quindi l'impegno al Governo di attivare ogni possibile canale per acquistare al di fuori di quello

che abbiamo definito tale in Commissione, nel testo peraltro ottimamente elaborato dalla Presidente,

paradossalmente potremmo essere pronti, se solo avessimo la disponibilità dei vaccini, e di questo evidentemente ci stiamo preoccupando un po' tutti. Sostanzialmente io manifesto, in questo ultimo lasso di tempo che mi è concesso, la soddisfazione per essere arrivati a redigere un documento unitario anche sulla campagna vaccinale, il che non era affatto scontato.

rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, stiamo affrontando il momento più difficile dall'inizio di questa emergenza sanitaria che si è presto trasformata in una emergenza sociale ed educativa, oltre che economica. Il Paese è provato da più di un anno di restrizioni, purtroppo necessarie per tutelare la salute dei cittadini e, nonostante il traguardo appaia meno lontano, la tenuta sociale e quella psicologica sono a rischio. Oggi siamo tutti consapevoli che i vaccini e la possibilità di coprire nel minor tempo possibile la maggior parte della popolazione, a partire dai più anziani e dai più fragili, costituiscono l'elemento decisivo per raggiungere in tempi celeri l'immunità di gregge e per superare questa drammatica emergenza. La ripresa passa attraverso l'efficacia e la velocità della campagna vaccinale con cui si abbattono le curve dei contagi, dei ricoveri, dei decessi. La scienza e la ricerca hanno messo a disposizione dei Governi più di un vaccino sicuro ed efficace in meno di un anno, a dimostrazione di quanto sia importante promuovere investimenti in sviluppo e ricerca nel settore scientifico sanitario. È evidente che è stata altresì fondamentale la scelta europea di una strategia comune, di una regia unica negli acquisti, ma non possiamo ignorare che sono stati commessi errori nella negoziazione contrattuale e nel rafforzamento della capacità produttiva industriale. Non è un caso che ora si stia correndo ai ripari su entrambe le questioni, con l'*ultimatum* dell'Unione europea dell'Unione europea ad AstraZeneca per colmare i ritardi nelle forniture di dosi concordate. Da questo punto di vista ci siamo preoccupati con ritardo anche del tema della capacità produttiva delle aziende che hanno realizzato i vaccini. Sarà un monito per il futuro, ma oggi non è il tempo di soffermarci sui possibili errori; è il momento di mettere in campo tutte le nostre energie per ottenere un risultato vitale per l'Europa e per il nostro Paese: quello di non arrivare in ritardo al raggiungimento della immunità. Per riuscire nell'intento dobbiamo superare innanzitutto le disparità territoriali, con cui spesso è stata gestita la campagna vaccinale. In questo senso accogliamo con soddisfazione l'ordinanza con cui il commissario Figliuolo ha indicato alle Regioni le priorità vaccinali per gli *over* 80 e le persone vulnerabili. Le linee guida contenute nel piano vaccinale non sono state un elemento sufficiente per molte Regioni per comportarsi in modo virtuoso, razionale, lungimirante. Adesso dobbiamo guardare al futuro e procedere alla vaccinazione di coloro che, in base alle evidenze scientifiche, corrono i rischi maggiori se contraggono la malattia, ossia mettere in sicurezza le persone anziane, in cui si concentra più del 95 per cento dei decessi, e coloro che hanno note di particolare fragilità per la loro condizione. Storie di morte e solitudine ce ne sono state tante e la qualità della democrazia di un Paese e della sua civiltà si misura proprio sulla capacità di tutelare e proteggere i più fragili. Devo dire con dispiacere il federalismo sanitario ha mostrato certamente qualche esempio virtuoso ma anche dei limiti, determinando discriminazioni, mentre la salute è un diritto costituzionalmente garantito che non prevede differenze, deroghe o salti di fila. Il sistema sanitario come bene comune vale per i cittadini come vale per tutte le prestazioni erogate, che hanno subito un inevitabile arresto con l'impennata della crisi. Corriamo il serio rischio che, usciti dall'emergenza Covid, la situazione subisca contraccolpi ulteriori e non possiamo permetterlo, perché il nostro sistema universalistico va difeso, perché è valutato come uno dei migliori al mondo. Su questo tema dobbiamo essere uniti. Sulla questione di cui tanto si parla e che riguarda gli eventuali rischi legati alla somministrazione del vaccino AstraZeneca, ritengo siano stati commessi degli errori di comunicazione, ma che sia necessaria una immediata campagna informativa che tranquillizzi i cittadini. Temo che inseguire il consenso pubblico nell'impossibile tentativo di promettere un rischio zero sia una strada fuorviante, perché si fonda su una motivazione solo politica e non scientifica. Ora il pericolo più grande che corriamo è che cresca la sfiducia dei cittadini nei vaccini e nelle istituzioni. C'è infine un tema che mi sta particolarmente a cuore, perché riguarda la mia città e ha a che fare con la civiltà del diritto. Nelle nostre carceri, e in particolare nell'istituto penitenziario di Reggio Emilia, starebbe aumentando in modo significativo la concentrazione di positivi, con il rischio di sommosse e disordini. C'è un'emergenza che riguarda la vita delle persone e, se non si è in grado di provare solidarietà per chi sta scontando una pena, almeno si provi ad averla per i lavoratori impegnati nelle strutture penitenziarie, luoghi chiusi per definizione e sovraffollati. Per questo sarebbe importante riflettere sulla possibilità di andare avanti sulla somministrazione dei vaccini ai detenuti e alle guardie carcerarie. Si tratta infatti di comunità in perenne emergenza. Colleghi, anche quando la fase acuta dell'emergenza - come speriamo - potrà essere attenuata e la campagna vaccinale avrà sortito gli effetti benefici auspicati, sarà necessario aver costruito una rete di protezione, perché il Covid, con le sue varianti, non scomparirà nel breve periodo. Occorrono una rete di protezione che preveda un piano nazionale di sorveglianza attiva, con uno *screening* diffuso e gratuito della popolazione. La chiusura delle agenzie educative ha prodotto danni gravi dal punto di vista degli apprendimenti, ma anche sul versante educativo e psicologico vi sono criticità che lasciano sconcertati. Occorre una rete di protezione che si fondi su altri strumenti diagnostici Covid e un piano di monitoraggio per bloccare, con misure tempestive, le varianti, scongiurando il rischio di inefficacia dei vaccini; una rete che si fondi sul rafforzamento delle cure domiciliari e della medicina territoriale. Nel frattempo, dobbiamo impedire che la campagna vaccinale subisca altre brusche frenate, che sarebbero molto gravi e, per farlo, serve una comunicazione delle istituzioni e della comunità scientifica chiara, che si esprima in modo semplice, spiegando le ragioni che motivano ogni scelta, rassicurando i cittadini. Serve una migliore strategia di approvvigionamento delle dosi. Ora, nell'annunciare il voto favorevole del PD, voglio soffermarmi sul concetto di resilienza, un termine molto usato negli ultimi tempi. La resilienza, dal latino *resilire*, è non solo di resistere, ma anche di risalire, di affrontare e superare le avversità. L'intelligenza e la forza di una comunità direttamente proporzionali alla sua capacità di affrontare le criticità di un sistema che muta, traducendole in opportunità. Invito dunque ognuno di noi a interpretare questo drammatico passaggio della storia del Paese nella direzione di una rinascita, di una ripartenza che potrebbe darci maggiori opportunità a patto che, nei prossimi mesi, sappiamo remare tutti nella medesima direzione.

che si sta svolgendo in questi giorni sul tema delle riaperture. Il nostro Paese è stanco, i cittadini italiani sono stanchi e preoccupati e sono tante le manifestazioni in atto, ma la risposta più seria da parte nostra alla tensione non è certo quella di cavalcarla. Il Paese ha bisogno di definire una prospettiva e un percorso chiari, ma certamente le strumentalità nei confronti del ministro Speranza non andranno da nessuna parte. ben risposto il presidente del Consiglio Draghi, si può e si deve aprire, costruendo un percorso in sicurezza e lavorando su tre livelli insieme: vaccinazione, tracciamento e tamponi. Solo così possiamo riaprire le

Finché non saremo capaci di riattivare il tracciamento collegato ai tamponi, riaprire è un percorso complesso. Dobbiamo dirlo con onestà e con chiarezza ai cittadini. Ieri abbiamo fatto un incontro con un'associazione di ristoratori e di gestori di palestre. Credo che questo ragionamento siano in grado di capirlo, se la politica, il Governo, le istituzioni insieme e la Repubblica sono capaci di pronunciare parole chiare, sincere e oneste rispetto al percorso che ancora dobbiamo

chi si muove diversamente deve vedere un intervento del Governo, perché nessuno

A tal proposito, si pone un grande problema. Come assicuriamo, in questa campagna e per il futuro, che i vaccini siano a disposizione come bene comune per tutti i cittadini? E mi riferisco a tutti i cittadini del mondo,

Fino a che, come previsto dagli accordi Trips, non si è data la possibilità di produrre i farmaci per l'AIDS al Sudafrica e ad altri Paesi in grande difficoltà,

non credo che questa sia la comunicazione più giusta per dare certezza ai cittadini. Occorre forse invertire il meccanismo, rassicurando lanciando messaggi tipo quelli che abbiamo dato sul numero dei vaccini che arrivano,

alla salute e alla vita delle persone, Forza Italia ha sempre dato - anche dall'opposizione, nei precedenti Governi - quel supporto istituzionale utile a fare squadra per il Paese per superare l'emergenza sanitaria. abbiamo proposto in quest'Aula, con la guida del capogruppo Anna Maria Bernini, delle soluzioni tecniche e sanitarie che poi sono state considerate valide e opportune anche dal Comitato tecnico-scientifico. abbiamo proposto soluzioni e metodi per anticipare il virus ed evitare la diffusione veloce dei contagi. Oggi, con lo stesso spirito costruttivo di allora e con la responsabilità istituzionale di sempre, siamo impegnati ad attuare tutte le soluzioni possibili per far uscire il Paese il prima possibile dalla morsa pandemica. Tra le diverse proposte di Forza Italia, abbiamo elaborato e presentato al Governo Draghi il piano vaccinale, sul quale ho avuto l'onore e il privilegio di aver lavorato di aver lavorato personalmente come medico, insieme ai colleghi di partito di Forza Italia, e che il commissario Figliuolo ha apprezzato e condiviso in parte, con lo scopo unico di arrivare all'obiettivo dell'immunità di gregge il prima possibile. Abbiamo proposto e ottenuto la vaccinazione nelle farmacie, per permettere una possibile inoculazione del vaccino in modo più capillare. Abbiamo chiesto lo scudo penale per i vaccinatori, per incentivare tutti i medici e gli operatori sanitari a rendersi disponibili per inoculare i vaccini, perché per uscire dalla crisi serve vaccinare il più velocemente possibile tutti e in tempo breve. Sempre in materia di vaccini, colleghi senatori, aggiungo che oggi abbiamo depositato un'interrogazione al Ministro della salute per sapere a chi verrà attribuita la responsabilità qualora non vengano consegnati i vaccini nei termini e nei tempi prestabiliti, provocando ritardi nel raggiungimento dell'immunità di gregge ed aggravando così la crisi economica e finanziaria del nostro Paese, delle piccole e medie imprese e delle singole famiglie. Inoltre, con l'interrogazione abbiamo chiesto di conoscere chi risponde dei casi, rarissimi, di eventuali e gravi effetti collaterali. Anche qualora si verificasse un caso ogni 100 milioni di vaccinati, va comunque tenuto in considerazione per non lasciare sola quella famiglia che ha subito un grave danno da vaccino, e nello stesso momento per incoraggiare, per trasparenza amministrativa - è l'aspetto più importante - i cittadini a credere e avere fiducia nel grande lavoro che insieme stiamo portando avanti, convintamente, sul piano vaccinale. Questo ci permette anche di superare la diffidenza verso alcuni vaccini; ne stiamo discutendo tutti i giorni in Commissione salute con il presidente Parente. Come ha denunciato il governatore Musumeci, in Sicilia l'80 per cento dei cittadini rifiuta il vaccino Astrazeneca. Questa oggi rischia di interessare, ingiustamente, anche Johnson & Johnson, secondo le notizie delle ultime ore. Ci sono grossi rallentamenti legati alla carenza di personale medico, soprattutto nelle Regioni commissariate come la Calabria. le società interinali contrattualizzate dal Governo non hanno contattato i medici in pensione che hanno già dato la loro disponibilità a vaccinare sin da subito. Ed è per questo che abbiamo fatto un ulteriore sollecito e abbiamo voluto che venisse inserito anche questo tema nell'ordine del giorno presentato. Non è condivisibile il fatto

Anche all'interno della mia categoria, quella dei medici, riscontriamo la denuncia di alcuni colleghi che non si sono vaccinati e che addirittura sbagliano - mi permetto di dirlo in quest'Aula ai colleghi - perché sconsigliano di vaccinare: questo è il più grande errore. Per altro verso, bisogna fare presto e bene per dare risposta a quella parte del Paese che scende giustamente in piazza per chiedere al Governo di fare presto, di fare il prima possibile in quanto la crisi sta schiacciando le famiglie italiane e le piccole imprese che temono di non farcela più per ripartire. Tutto il nostro partito, con il presidente Berlusconi e il vice presidente Tajani, ha chiesto al Governo di fare una verifica della situazione il 20 aprile, per valutare - naturalmente seguendo i parametri tecnici, tra i quali la curva del contagio e l'attuazione del piano pandemico - dove è possibile riaprire le attività. per questa ragione stiamo lavorando per presentare al presidente Draghi un piano tecnico per favorire le riaperture in sicurezza e il prima possibile.

Tuttavia, è arrivato il momento di cambiare passo e accelerare decisamente verso il traguardo finale. A nome del Gruppo parlamentare Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC annuncio il voto favorevole all'ordine del giorno unitario, in quanto contiene una relazione dettagliata, compiuta e completa della situazione vaccinale odierna e contribuisce politicamente a dare soluzioni per velocizzare e rendere più efficiente piano vaccinale accogliendo le nostre proposte. L'ordine del giorno, in effetti, tra i tanti punti affrontati, impegna in particolar modo il Governo con urgenza a rivedere il piano vaccinale per superare i ritardi attuali, attuali, nel senso di accoppiare i tipi vaccinali adeguati ai *target* di età, potenziando le risorse umane sanitarie impegnate nella vaccinazione. Inserisce, altresì, tra le priorità vaccinali coloro che operano a contatto con il pubblico e, tra questi, anche il personale docente e non docente della scuola; prevede di reprimere e sopprimere gli eventuali abusi, come per esempio il famoso elenco di cittadini vaccinati che si trovano sotto la voce "altro" - giustamente rilevato anche dal presidente Draghi - dove si possono leggere i nomi di coloro

e impegnare adeguate risorse, sia nel campo della ricerca, degli anticorpi monoclonali, del vaccino italiano ReiThera, sia sulla valutazione dei *follow-up* delle persone vaccinate, fondamentali per capire cosa accadrà nei prossimi mesi rispetto al piano vaccinale che stiamo attuando, convinti che è l'unica arma per poter uscire dalla pandemia. Il nostro è quindi un convinto sì all'ordine del giorno e un pieno appoggio al Governo, perché riesca a tradurre in azioni concrete gli elementi che il Parlamento gli affida del Governo, che, accogliendo la nostra proposta sul piano vaccinale, si esalta il significato del vaccino, inteso come strumento che azzera le disuguaglianze nel mondo, colorando di luce e di speranza il diritto alla salute, che diventa veramente universale alla portata di tutti i cittadini del mondo e, nello stesso tempo, uno strumento di solidarietà perché ci si vaccina non soltanto per se stessi, ma soprattutto per prevenire la trasmissione del virus

posto che sono già stati fatti molti interventi di pregio sull'argomento, assorbenti quanto avrei voluto esporvi, vorrei solo sottolineare, come ebbi già avuto modo di dire anche in quest'Aula, che non sono i vaccinatori a mancare, ma i vaccini. Quindi, ben venga tutta l'attenzione al reperimento delle dosi, com'è stato annunciato e secondo gli impegni dedotti nell'ordine del giorno. Mi raccomando anche di dare la giusta attenzione alla previsione del piano di sorveglianza attiva e genomica, di governo della mutabilità del virus, di contenimento in sicurezza nelle sue varianti e di monitoraggio delle loro interazioni con il sistema immunitario e con i farmaci, a garanzia dell'immunizzazione di massa. Chiunque abbia idee pratiche su come approvvigionare quantitativi addizionali in emergenza merita di essere supportato, purché iniziative coerenti con il quadro di riferimento europeo. Approfitterei dei pochi minuti restanti per invitarvi ad una stravagante quanto paradossale riflessione, che potrebbe suonare più o meno così: «Benvenuto Covid». Se è vero, infatti, che abbiamo avuto 115.000 vittime per la pandemia, altrettanto vero è che, in modo miracolistico, dalle statistiche ufficiali pare che siano 'scomparsi' i morti per infarto, per cancro e altre patologie, almeno nei mesi di gennaio e di febbraio di quest'anno. Ho cercato infatti di confrontare i dati rilasciati dall'Istat sui decessi ufficiali e, non da sola per la verità, ci siamo resi conto che c'è qualcosa che non quadra. L'Istat attesta, invero, che la mortalità a livello nazionale nei mesi di gennaio e di febbraio è marginalmente superiore a quella della media degli anni precedenti. Ad uso esclusivo degli amanti dei numeri: 1.125 in più in due mesi, già depurati dei dati del 2020. Sempre tanti, perché di persone trattasi, ma, a differenza di quanto è successo a inizio pandemia, oggi non c'è quell'ecatombe che siamo abituati quotidianamente ad ascoltare e che ci dà conto di una media giornaliera ponderata di oltre 400 decessi Covid; se così fosse, in due mesi sarebbero pari a circa 24.000 decessi in più, rispetto ai 1.125 registrati, e dovrebbero trovare contezza nelle statistiche. I vaccini sicuramente hanno contribuito al calo della mortalità, perché, seppur a macchia di leopardo e con qualche inefficienza, nello stesso periodo sono stati 4 milioni quelli che hanno avuto almeno la prima dose, il che senz'altro ha contribuito a contrastare la diffusione del Covid. Ma ciò non basta a spiegare questa discrasia. Sono certa che ci sarà un momento in cui sarà fatta luce anche su questo nel frattempo, essendo state profuse tutte le energie necessarie sui vaccini è sicuramente in grado di arrivare a 500.000 vaccinazioni giornaliere, penso che sia nostro dovere tutelare coloro che sono affetti da altre patologie, che a causa del Covid sono state depriorizzate. nella trattazione della precedente mozione, non è possibile che su tutto il territorio nazionale, nei mesi di gennaio e di febbraio, i morti per le prime dieci patologie che affliggono la nostra società siano diminuiti di oltre 22.000 unità,

Se così fosse, ci dovremmo porre interrogativi ancor più gravi. Da qui nasce la mia 'stravagante' riflessione "se il Covid faccia guarire da tutte le altre patologie": siccome questo non è vero, sarà necessario fare luce sul perché in Italia risultano rilevati molti più morti per Covid che negli altri Paesi dove la sanità è uguale o anche meno efficiente della nostra. questo l'abbiamo già visto - nonostante la mancanza del piano pandemico e il mancato massiccio ricorso alle cure territoriali, ci sia stata da una parte una spropositata conta di decessi (esclusi i primi due mesi, quando si brancolava nel buio) e dall'altra una miracolistica guarigione immotivata. Invito a riflettere, ma contestualmente ad andare oltre, non facendo mancare il nostro supporto al sistema, per intervenire in modo tempestivo e appropriato sulle vaccinazioni, sì da poter dedicare tutte le attenzioni verso le altre patologie. Questo dovrebbe essere il senso ultimo dell'ordine del giorno che ci apprestiamo ad approvare, al di là degli specifici impegni richiesti al Governo per una profilassi vaccinale che sia così capillare e diffusa da evitare altre successive recrudescenze: coniugare piano strategico vaccinale e piano nazionale di recupero delle attività di *screening*, di presa in carico e degli interventi

prendo la parola in quest'Aula sempre più convinta che, al termine di questa emergenza sanitaria, sarà necessario aprire una seria riflessione sul Titolo V della Costituzione. L'autonomia regionale nella gestione della sanità ha mostrato tutti i suoi limiti e, come il MoVimento 5 Stelle chiede da anni, non sarà più rinviabile una discussione in merito. Sappiamo tutti benissimo che questa pandemia ha messo a dura prova il nostro Servizio sanitario nazionale, reduce da tagli che si sono perpetuati negli anni: circa 37 miliardi di euro in dieci anni. L'aspetto positivo è che anche chi di quei tagli è stato responsabile quando era al Governo sembra oggi aver finalmente capito che sulla sanità non si può lesinare. Abbiamo visto anche che alcuni sistemi regionali, quelli in cui - ad esempio - si era puntato molto sul privato, depauperando la medicina del territorio, hanno sofferto più degli altri; penso, per esempio, alla Lombardia. Abbiamo visto Regioni che, pur di non abbandonare i propri sistemi di prenotazione regionale in favore di quello statale di Poste Italiane, sono andate incontro a problemi gravissimi. Abbiamo visto e purtroppo vediamo ancora differenze regionali sia nella campagna vaccinale che nell'uso dei monoclonali: Regioni in cui si è scelto di dare precedenza ad alcune categorie professionali anziché agli anziani (guardiamo l'Umbria con gli avvocati); Regioni in cui gli anticorpi monoclonali sono stati consegnati, ma non sono stati usati (eppure sappiamo benissimo che si tratta di una terapia in grado di ridurre in modo drastico un decorso nefasto della malattia e i ricoveri in terapia intensiva); in Calabria è stato trattato un solo paziente. Abbiamo poi visto *boutade* elettorali, come quella fatta dal governatore De Luca, che non vuole dare precedenza ad anziani e fragili, peraltro sconfessando quanto deciso in Conferenza Stato-Regioni. Come se non bastasse, assistiamo a una diatriba sulle riaperture, quasi si trattasse di una presa di posizione politica, una specie di finto braccio di ferro tra "aperturisti" e "rigoristi", con date lanciate a casaccio, che alimentano le ansie dei cittadini, quando basterebbe davvero un po' di senso di responsabilità; lavorare sui ristori, come abbiamo fatto fino ad ora; ragionare sulle riaperture in modo laico, trattandosi di una questione sanitaria, partendo dai dati scientifici e dall'andamento della campagna vaccinale. In tutto questo abbiamo dei punti fermi. Sappiamo per esempio - o dovremmo saperlo tutti che le fasce a zone sono quelle che ci hanno consentito negli ultimi mesi di fare delle riaperture e che in questo anche l'andamento della campagna vaccinale gioca un suo ruolo. È imprescindibile procedere sulla base dell'età e del rischio medico, perché solo mettendo in sicurezza chi rischia conseguenze più gravi potremmo avviarci all'apertura in sicurezza. Proteggiamo i più fragili: in questo modo arriveremo ad avere meno ricoveri in terapia intensiva, gli ospedali soffriranno meno e riusciremo a riaprire. Non c'è spazio, certo, per quella scelta scellerata di illudere chi ha pagato le conseguenze peggiori delle chiusure. È tremendo scegliere di far leva su questo per racimolare dei voti. È tremendo prendere in giro i cittadini; dobbiamo essere sinceri: meglio attendere una settimana in più prima di aprire, ma farlo in sicurezza. Evitiamo il ripetersi di quanto accaduto con la Sardegna che, dopo due settimane di liberi tutti, è ripiombata prima in zona arancione e ora addirittura in zona rossa. Allora, da un lato i vaccini e dall'altro i ristori. Sul fronte dei vaccini non si può sottacere un atteggiamento vergognoso da parte di alcune case farmaceutiche che ritardano le consegne e alzano i prezzi. Per questo il MoVimento 5 Stelle sta portando avanti una battaglia ben precisa. Dobbiamo attrezzarci per la produzione locale, soprattutto di vaccini a mRNA e dobbiamo liberalizzare i brevetti con gli strumenti consentiti dai accordi Trips. È fondamentale sia per velocizzare la campagna vaccinale sia soprattutto per garantire che i vaccini arrivino a tutti, anche ai Paesi più poveri. Non sfugge a nessuno che da questa pandemia è il mondo intero a dover uscire, e non solo una parte, non solo la parte ricca che si può permettere i vaccini, ma tutti quanti; è un discorso etico, un discorso di sicurezza sanitaria. In tutto questo è importante non abbandonare l'azione globale portata avanti dall'Europa. Da quel *vaccine day* del 27 dicembre sono successe molte cose, ma ci sentiamo di scongiurare in ogni modo la spinta all'uso di vaccini non approvati dall'Agenzia europea dei medicinali. Basti guardare cosa sta accadendo, per esempio, in Cile, dove la politica ha deciso al posto della scienza: hanno usato un vaccino che non era stato testato a sufficienza e ora si ritrovano con i contagi in salita e con una copertura non sufficiente della popolazione. modo, non possiamo rivolgerci ai mercati paralleli, come propone qualche Presidente di Regione, che non forniscono garanzie e possono alla fine risultare penalizzanti per la strategia comune europea. Ci sono stati intoppi - è inutile negarlo - ma non dobbiamo nemmeno dimenticare che è grazie ai vaccini se riusciremo a lasciarci alle spalle questa pandemia. E allora muoviamoci per risolvere le criticità: sospendiamo le licenze, iniziamo a produrre i vaccini, iniziamo a non dover più dipendere da nessuno; un piccolo passo per riprenderci quanto abbiamo di più caro nel modo più veloce possibile: la nostra libertà. Per questo, il voto del MoVimento 5 Stelle sarà favorevole all'ordine del giorno unitario. *(Applausi)*.

di merito e di metodo: di metodo, perché l'ordine del giorno è pervenuto pochi minuti fa e, quindi, non ci ha consentito una disamina approfondita; di merito, perché basta leggere il primo capoverso per vedere una narrazione autoassolutoria di tutti i partiti che compongono la maggioranza e anche la finta opposizione. Basti leggere che «il sistema nazionale ha risposto nel miglior modo possibile»: non è vero. La realtà è assolutamente diversa... *(Commenti).* PRESIDENTE.

senatore. CRUCIOLI *(Misto)*. Ci sono stati errori evidenti sia nel reperimento dei vaccini sia nella scelta delle persone da vaccinare, come nelle chiusure che sono state eccessive. Adesso qui si dice che invece il sistema ha risposto nel miglior modo possibile. Non è vero. Voteremo contro. L'Alternativa C'è è l'unica opposizione.

non stiamo attribuendo un'eccessiva rilevanza? Indìco

Comunico che la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, di cui alla mozione approvata dall'Assemblea del Senato il 30 ottobre 2019, è stata convocata, per la sua costituzione, giovedì 15 aprile 2021, alle ore 12,30, nell'Aula della 10a Commissione permanente. **Atti